Ma perché non chiede scusa, senatore Garraffa, per i suoi comportamenti, quando è intrinsecamente così? Ma cerchi di essere normale! È una prassi consolidata da parte di tutte le Presidenze, di destra e di sinistra, di tutte le maggioranze, che per il primo voto c'è tolleranza

come i colleghi sanno visto che ieri se ne è discusso molto in quest'Aula, e se ne era discusso, peraltro, anche in sede di Conferenza dei Capigruppo, noi avevamo chiesto che alla seduta di oggi presenziasse il Presidente del Consiglio, onorevole Berlusconi. Notiamo invece la sua assenza e la presenza, che ci è sempre gradita, naturalmente, del ministro Alfano. La nostra richiesta non era rivolta alla possibilità o alla fortuna di avere un oggetto di contemplazione (in questo caso un soggetto di contemplazione, cioè il Presidente del Consiglio),

sapere da parte del Governo, che in maniera del tutto inconsueta pone la questione di fiducia su un testo di schietta origine parlamentare senza neanche curarsi - lasciatemelo dire - di coprire la

di legislatura che vengono originati da libere elezioni, nel momento in cui il Governo investe le Camere di un voto di fiducia su un oggetto specifico, vuol dire che ritiene quell'oggetto specifico meritevole meritevole della prova di responsabilità che è il voto di fiducia, lo assume cioè come punto prioritario del proprio programma, come condizione essenziale per continuare nell'esercizio dell'attività di Governo.

e che contiene norme sul legittimo impedimento, considerandole priorità dell'azione di governo, nel momento in cui - lo ripeto - il Paese sta marcendo per ragioni diverse e una grande questione economica, sociale, democratica si apre nel Paese. del senatore Li Gotti).* Vorrei, a nome del mio Gruppo e immagino anche a nome degli altri colleghi dell'opposizione, che a questa domanda venisse data risposta dal ministro Alfano, il quale è oggi qui in piena rappresentanza del Governo nell'assenza del presidente Berlusconi che, visto che il provvedimento peraltro è fatto per lui, avrebbe potuto avere la cortesia istituzionale di scomodarsi e di presenziare ai nostri lavori.

preferisca non essere in quest'Aula per affrontare un tema così delicato. Le chiediamo dunque, Presidente, di informarci sulla presenza o meno del presidente Berlusconi. Ministro per i rapporti con il Parlamento allo stato attuale non mi ha dato conferma della presenza del Presidente del Consiglio, mentre prendo atto della presenza del ministro Alfano, che era stata anch'essa invocata da alcuni Gruppi, seppure in aggiunta a quella del Presidente del Consiglio. Non posso che prendere atto di questo stato di cose e, dunque, della presenza del Ministro della giustizia. Come ho ribadito ieri, non esistono strumenti e mezzi in capo al Presidente del Senato per imporre al Presidente del Consiglio di essere presente in Aula.

La presenza del ministro Alfano è un *quid pluris*, un fatto in più rispetto allo scenario di ieri, in cui il Governo era rappresentato solo dal sottosegretario Alberti

abbiamo alle spalle due anni di legislatura e i problemi della giustizia restano centrali: credo che nessuno possa contestare la centralità dei problemi della giustizia. Ebbene, a fronte di una crisi devastante riguardante l'organizzazione giudiziaria ed il servizio giustizia, vi chiedo: cosa si fa in un Paese civile? Prima di rispondere a questa semplice domanda, intendo chiarire cosa ritengo sia per me un Paese civile. Si tratta di un Paese dove prima di ogni altra riconosciuto un doveroso e profondo rispetto verso la legge, la cui centralità e, direi anche sacertà, ha alle spalle ormai due millenni

con procedura d'urgenza (che a voi è così cara), in modo concordato (ve ne erano i presupposti, davanti alle nostre proposte di legge, all'inizio della legislatura) alcune di queste norme che contengono gli strumenti di riforma strutturale affinché si potessero risolvere i problemi della giustizia.

questa storiella, questa leggenda dei giudici italiani persecutori. Sottolineo con molta schiettezza che il numero elevato dei coinvolgimenti giudiziari del Presidente del Consiglio dei ministri dipende esclusivamente dalla sua storia, dal suo tenore di vita.

che comincia a diventare veramente pesante e difficile da accettare. Questa è una prerogativa, ha bisogno di una procedura di riforma costituzionale: lo ha detto la Corte; lo sapete anche voi. Avete dato la prova di questa percezione, di questa sensibilità - se così si può definire - quando, paradossalmente, nel disegno di legge avete inserito una previsione di una successiva riforma successiva riforma costituzionale, quasi a dire: «Noi adesso variamo questa legge d'urgenza, poi metteremo le cose a posto». Ora però spiegateci - perché questo vuole la legge - in modo civile e rispettoso le ragioni per cui voi ponete la questione È questo un istituto previsto dalle norme vigenti che presuppone evidentemente ragioni politiche rilevanti, perché altrimenti il sistema legislativo democratico ne risente in modo grave. In modo particolare, In modo particolare, si pone la questione di fiducia quando si intravede un contrasto interno, quando vi è un possibile pericolo che nella maggioranza vi siano cedimenti o punti di vista differenti o vi sia un'insufficienza numerica. Parlo del Governo Prodi: voi rinfacciate che in quella fase noi abbiamo dovuto ricorrere all'istituto della fiducia, ma in quel caso si spiega, vi è una ragione politica valida. Oppure - e qui vi richiamo all'attenzione e alla riflessione, e mi rivolgo in particolare al ministro Alfano - vi deve essere un pericolo di ritardo nel varo delle riforme, relativamente al valore o all'interesse che le norme in esame vogliono tutelare. Ministro Alfano, ci spieghi qual è il valore o l'interesse che queste norme intendono tutelare e qual è il pericolo nel ritardo. Ieri il Vice Presidente del Gruppo di maggioranza,

L'arroganza viene vista addirittura nell'esercizio sacrosanto del diritto‑dovere dell'opposizione di rispondere a leggi e a comportamenti, quelli sì arroganti, con una serie di emendamenti che sono stati studiati, sofferti e presentati nella legittima aspettativa di poterli discutere con voi. Vi chiedo allora: poiché avete una maggioranza così netta e schiacciante, cosa vi spaventa? Anche il confronto con un'opposizione che finora ha dato e darà sempre prova di civiltà, di compostezza e di coerenza con le norme, la legge (amici e colleghi della maggioranza:,questa parola che vi fa tanta paura e vi disturba)? Il nostro è un atteggiamento di opposizione duro, netto nei confronti di un comportamento della maggioranza che sta scivolando verso un sistema che, non rispettando la legge, potrebbe essere il prodromo di uno scivolamento verso un regime. Questo sembra lasciarvi assolutamente insensibili ed è proprio questo che preoccupa i veri democratici.

per la verità devo complimentarmi con il ministro Alfano per essere venuto in Aula, perché in fin dei conti anche la questione è un atto del Consiglio dei ministri. Ho visto che oggi diversi Ministri sono presenti in quest'Aula e me ne compiaccio.

Furono varate senza ricorrere, all'inizio, a leggi costituzionali perché non era necessario. Fu fatta la legge sulle rogatorie: si pretese che le rogatorie fossero autenticate. Allora facevo ancora il magistrato e ricordo che, effettivamente, quando chiedemmo

E fu la prima legge, in sostanza disapplicata, che non servì agli scopi. Poi si fece la legge sul falso in bilancio, in un momento in cui

del Presidente del Consiglio. Credo che la ragione per cui ci troviamo tutti quanti a discutere sia la legge costituzionale n. 3 del 29 ottobre 1993 che abolì l'autorizzazione a procedere. Probabilmente non ci saremmo dovuti trovare tutti qui a discutere:

non vorrei che anche per questa legge succedesse quel che è successo per le altre leggi fatte in precedenza con lo stesso intento.

a Milano, si portasse questa legge approvata - e forse la fiducia è stata messa proprio per questa ragione - e poi si dicesse: i soliti magistrati sovversivi hanno presentato di nuovo la questione di legittimità costituzionale e hanno mandato la legge davanti alla Corte costituzionale. Si è parlato di legge ponte, temporanea, ma forse non c'era neanche bisogno di farlo, perché anche il lodo Alfano valeva per un certo tempo, fino a che la Corte costituzionale non l'ha poi dichiarato illegittimo, i suoi effetti li ha prodotti, tant'è vero che il processo è stato sospeso. Per la verità, quando mi telefonarono e mi dissero che era stato assolto Mills mi sentii quasi sollevato: vuoi vedere che adesso veramente ci occupiamo dei problemi del Paese anziché dei problemi del Presidente del Consiglio? Perché questa è la storia. Noi ci troviamo in un momento difficilissimo del nostro Paese, nostro Paese, in cui l'economia va a rotoli, in cui bisognerebbe pensare effettivamente a rilanciare l'economia e l'occupazione: invece qui al Senato ci occupiamo di questi problemi. Fin dal 2005, signor Ministro, proposi che si risolvesse il problema della conflittualità, così come viene chiamata, fra magistratura e mondo politico. Non voglio riprendere i termini che ha usato il mio ex collega Davigo,

Così come andava risolto con l'accordo, e non con un decreto-legge, il problema relativo alle elezioni in Lombardia e nel Lazio. Volete la nostra collaborazione: ebbene,

Eugenio Scalfari lo ha scritto chiaramente: forse la soluzione migliore in questo momento per risolvere il problema della conflittualità è quella che è stata proposta da Gerardo D'Ambrosio.

va fatta con la procedura delle leggi costituzionali: quindi ci troveremo, tra poco, di nuovo di fronte a questo problema, ad un'altra dichiarazione di incostituzionalità. Poi, legge ponte: farete questa legge costituzionale, ma come ve la farete? Ve la farete da soli,

vedere se è efficace o no: come andrà a finire? Come vedete, quando invocate la collaborazione dell'opposizione non è un'invocazione vana, perché l'opposizione è necessaria, è indispensabile, per risolvere questi problemi. Se volete farne a meno, siamo qui; fatene a meno e andate avanti per la vostra strada, ma poi non lamentatevi quando interverrà la Corte costituzionale e vi dirà che anche questa legge non è costituzionale.

La motivazione deve essere: vi spiego qual è il rapporto tra l'urgenza di questo provvedimento e il programma del mio Governo, un rapporto così stretto al punto che metto in gioco la fiducia, cioè metto in gioco il Governo stesso su questa partita. Questo dovrebbe spiegarci il ministro Alfano. Il silenzio che viene dal banco della Presidenza mi fa capire che il mio punto di vista non è da questa condiviso: pazienza, non è la prima volta.

passaggio è particolarmente grave perché interviene su un atto del Parlamento, su un disegno di legge di iniziativa parlamentare e non del Governo, e non è nemmeno legato ad un maxiemendamento che avesse tentato in qualche modo di tener conto del dibattito e degli emendamenti presentati, nonché su un argomento che non è nel programma

pubblico, non si possono dire in un'Aula istituzionale. Questo Governo non può alzarsi e dire la verità, dire ai ragazzi che ci ascoltano: «Sì, questo provvedimento è urgente e noi poniamo la questione di fiducia; ci giochiamo la faccia, la nostra, del Governo, della continuità della legislatura, perché non vogliamo che il Presidente del Consiglio si faccia processare». Questa cosa non si può dire in un'Aula istituzionale, ma è la verità. Non possiamo andare avanti con questo dibattito come in una specie di fiera della falsità,

siamo abituati da questo centrodestra, soprattutto in questa legislatura, del *superior stabat lupus*, per cui il lupo rimprovera all'agnello di essere lui che provoca per farsi mangiare: questa è la tecnica

ricordo solo che avevamo fatto delle aperture sulle riforme istituzionali, ma anche che avessimo parlato di tale questione

è lo strumento, di cui non riusciamo a capire il senso. Mi permetto di dire che l'unico strumento possibile in una democrazia civile è è il processo breve *ad personam*. Dovremmo cioè avere un provvedimento secondo il quale il Presidente del Consiglio per esercitare serenamente - visto che abbiamo introdotto questa nuova categoria politico-giuridica della serenità del Presidente del Consiglio Presidente del Consiglio - il suo mandato, avendo delle pendenze con la magistratura, vuole essere processato in 15 giorni, in fretta, passando davanti a tutti, con procedure d'urgenza, perché la priorità per il Paese è togliere qualsiasi ombra dal Presidente del Consiglio. Allora noi ci stiamo a fare un ragionamento di questo genere, perché il bene prezioso non è la serenità del Presidente di poter governare senza l'intralcio fastidioso di doversi presentare ai processi; il bene prezioso è la serenità di tutti i cittadini italiani di potersi svegliare la mattina, andare a lavorare, avere la preoccupazione di far tornare i conti della giornata, portare i figli a scuola, affrontare tutti i mille problemi della vita quotidiana, sapendo di essere governati da una persona per bene,

tutti gli strumenti che democraticamente possiamo usare per opporci, un provvedimento che dice che per sei mesi e poi ancora per sei mesi e poi ancora per altri sei mesi il Presidente del Consiglio può non sottoporsi a giudizio. perché poi abbiamo pronto un altro provvedimento? Anche in merito a ciò non sono d'accordo, ma chi era d'accordo che questo potesse costituire un *escamotage*

quindi un Governo che vuole giocare quattro carte (è un gioco nuovo, non quello delle tre carte) e tenerle tutte sul tavolo per ricattare il Parlamento ed il Paese. Mi spiace usare parole grosse ma di questo si tratta, di un ricatto al Parlamento ed al Paese, della serie: finché non si passa questo guado qui non si discutono più i problemi della gente, qui non si fa più sul serio, non si fa più politica, perché questo è il guado che va passato.

per questa istituzione, dove ho l'onore di essere stata mandata dai cittadini italiani, per fare quello che invece facevano i colleghi del centrodestra. Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento in esame è palesemente contrario ai principi generali dell'ordinamento e allo Stato di diritto. Mi soffermerò sugli aspetti più gravi dell'articolo 1. Tale situazione è resa più grave dalla scelta tirannica del Governo di troncare immoralmente il dibattito parlamentare con la questione di fiducia. Il provvedimento al nostro esame introduce nell'ordinamento, con legge ordinaria, prerogative giudiziarie connesse all'esercizio della funzione politica, conducenti ad una sospensione automatica del processo - per il Presidente del Consiglio dei ministri e per i Ministri senza alcuna possibilità di valutazione concreta, da parte del giudice, della effettiva sussistenza degli impedimenti dell'imputato caso per caso. introdurre prerogative di ordine costituzionale connesse all'esercizio della funzione di governo, che conducono ad un rinvio, peraltro reiterabile, del processo. Il fatto stesso di ricoprire la carica comprime lo spazio per una verifica oggettiva da parte del giudice della sussistenza dell'impedimento, che

ad esclusivo vantaggio di una ben precisa categoria di imputati, che dovrebbero trarre serenità non dal blocco dei processi bensì da una loro celere celebrazione. Anziché individuare, tipizzandoli rigidamente, gli impedimenti strettamente connessi all'esercizio dell'attività del Presidente del Consiglio e dei Ministri - come indicato espressamente dalla sentenza n. 262 del 2009 della Corte costituzionale - la norma in esame, all'articolo 1, comma 1, sancisce che costituisce legittimo impedimento per il Presidente del Consiglio dei ministri e per i Ministri «il concomitante esercizio di una o più delle attribuzioni previste da leggi e da regolamenti e, comunque, attribuzioni connesse alle relative attività preparatorie e consequenziali, nonché di ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di governo». In sostanza, qualsiasi atto legittima l'impedimento. Ancor di più, per effetto del richiamo ad una imprecisata coessenzialità, l'oscurità e la indeterminatezza del testo si configurano in un privilegio per la carica che riguarderebbe anche processi per reati comuni iniziati prima dell'assunzione della carica di Presidente del Consiglio. Nella sentenza n. 262 del 2009 la Corte costituzionale aveva precisato come fosse «irragionevole e sproporzionato», rispetto all'esigenza di tutela dei diritti degli imputati, la previsione

la previsione secondo cui «costituisce legittimo impedimento» l'esercizio di una funzione sancita «dal regolamento interno del Consiglio dei Ministri» vigente, comprese le successive modificazioni. poiché è il Consiglio dei ministri che definisce il proprio regolamento, il Consiglio dei ministri stesso - *pro futuro* - deciderà ciò che potrà determinare legittimo impedimento per il Presidente del Consiglio e per i Ministri: altro caso di conflitto di interessi. La coessenzialità di cui parla il comma 1 dell'articolo 1 e l'inserimento anche degli atti consequenziali alle attività tipiche del Presidente del Consiglio e dei Ministri sono elementi che inducono a ritenere che l'articolo 1, comma 1, contrasti contrasti clamorosamente con l'articolo 420-*ter* del codice di procedura penale, perché fa coincidere le ragioni dell'impedimento con la carica e non già con l'esercizio di specifiche attribuzioni, valutabili dal giudice di volta in volta, caso per caso. Il riferimento, inoltre, anche ad attività preparatorie e consequenziali rischia di esorbitare peraltro anche dalle attribuzioni tipiche della carica governativa. Questa analisi del solo comma 1 è sufficiente a dimostrare come la giornata di oggi rappresenti la morte dell'articolo 3 della Costituzione.

mancate posizioni da parte della minoranza tese ad offrire un contributo, che si potrebbe definire costruttivo, pur in presenza di un disegno di legge che ha un contenuto di una tale audacia che fa reagire non soltanto noi dell'opposizione, ma il mondo intero per quanto sia forte il forte il tentativo di conseguire un obiettivo attraverso strumenti che il nostro ordinamento costituzionale non prevede. Tuttavia, non sono mancati contributi, in Commissione e anche negli emendamenti, tesi a ridefinire la figura del legittimo impedimento. Infatti, rispetto alla categoria generale del legittimo impedimento, così com'è disciplinato dal codice odierno, nel trattare la condizione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri, si poteva anche considerare un ragionamento ed un'articolazione di questa figura che, tenuto conto dei compiti e delle funzioni,

il Presidente del Consiglio e i Ministri non possono sottoporsi ad alcun procedimento penale, non possono mai comparire in un giudizio penale, perché

elementi che possono giustificare l'assenza del Presidente del Consiglio e dei Ministri anche categorie indefinite ma vastissime, come le attività preparatorie alle riunioni del Consiglio dei ministri, quelle consequenziali, ossia le attività precedenti e

Inoltre, la Presidenza del Consiglio certifica la qualità di queste condizioni e sostanzialmente ne definisce il contenuto come legittimo a produrre il risultato che la legge mette in campo. sono fattispecie ampie ed una sostanziale autocertificazione, perché, pur essendo la Presidenza del Consiglio un'organizzazione amministrativa con una sua autonomia, è innegabile che l'agenda, il calendario, gli umori, gli impegni del Presidente del Consiglio finiscono per determinare i contenuti di questa attività. Come se non bastasse, vi è una categoria ulteriore, quella del sereno svolgimento delle funzioni attribuite dalla Costituzione. L'aggettivo turba, preoccupa, a parte il fatto che introduce anche in questo caso elementi di vaghezza e di genericità. Il nostro ordinamento prevede le normali funzioni, lo svolgimento costante delle funzioni, il regolare svolgimento delle funzioni attribuite a chi ha una responsabilità pubblica, ma mai l'aggettivo "sereno", che implica anche una condizione psicologica particolare, che - mi sembra di capire - potrebbe essere messa in campo. Da chi? Probabilmente non più da un esponente dell'apparato burocratico della Presidenza del Consiglio. Chi certifica chi la testimonia? Uno psicologo, una seduta psicoanalitica? Chi ci dice che, tra le altre cose, il Presidente del Consiglio non può andare in tribunale perché quella mattina non è sereno e perché un avviso di convocazione presso un giudice determina l'assenza della serenità? chi ha assunto questa iniziativa legislativa si sia preso una libertà e abbia un approccio disinvolto con i canoni e i princìpi del nostro ordinamento giuridico. giuridico. La maggioranza, se ritiene, deve percorrere la strada che anche questa mattina ribadiamo, quella normale, quella giusta, quella che si può fare nel nostro Paese, cioè mettere mano alla Costituzione e introdurre

quelli che amano i formalismi e cercano nella forma soluzioni politiche, ma perché

non è possibile che questo impedimento sia generico e attenga a tutte le violazioni di norme che il Presidente del Consiglio e i Ministri possono compiere. Noi siamo dell'avviso - lo abbiamo già detto - che questa prerogativa può essere al massimo circoscritta ai reati che si possono commettere in relazione alla funzione pubblica che viene svolta e giammai a qualsiasi forma di violazione che naturalmente introduce dubbi e perplessità, ancora una volta non formali ma sostanziali, che rischiano di far prendere un declino alla democrazia del nostro Paese, la quale ha già qualche problema

Presidente, signor Ministro, colleghi, un provvedimento e - fatto gravissimo - un voto di fiducia che lacerano ancora una volta il tessuto vitale della nostra democrazia. Non c'è Paese democratico, avanzato, di grande rilievo nel contesto internazionale che vive la nostra misera condizione. È vero, in qualche Paese è prevista una sorta di scudo per alcune alte cariche istituzionali; ma sono previsioni ordinamentali astratte, impersonali, spogliate da qualunque riferimento a un caso concreto su cui ‑ come in Italia nel caso del presidente Berlusconi - sono in corso dei processi. C'è una questione di fondo che caratterizza il vostro supino modo di agire dentro le istituzioni: mi riferisco al rapporto che le classi dirigenti devono avere con il potere. È vero che nei Paesi avanzati, con democrazie solide e mature, si sono avuti processi istituzionali che hanno spostato il peso decisionale verso gli Esecutivi. Ciò ha consentito di mantenere alta la capacità politica, di mantenere il primato e la sua stessa capacità competitiva con altri poteri, soprattutto economico-finanziari. Decidere. Decidere velocemente ha trovato spazio perché si sono mantenuti i famosi bilanciamenti, i bilanciamenti tra i poteri, e soprattutto si è esaltata la responsabilità politica che in molti casi è più severa e selettiva della stessa responsabilità penale. Insomma, al potere corrisponde la responsabilità; in sintesi: più potere, più responsabilità. Nel nostro Paese, signor Presidente, signor Ministro, si è scatenata un'altra relazione: più potere, più privilegi; più potere, più impunità. Sui privilegi e sulle impunità si fonda la legge sul legittimo impedimento. Molti nostri colleghi hanno svelato il carattere arbitrario, discrezionale, autoreferenziale a stabilire quando si è impegnati nell'azione di Governo: insomma, un'altra norma per stare fuori dai processi per avere un percorso fuori dalla giurisdizione costituzionale e universalmente poggiata sull'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, per di più se si è esponenti massimi delle istituzioni come il Capo di un Governo. Sulla giustizia, nel frattempo, niente. Niente sul processo telematico; niente sulle risorse finanziarie; neanche la possibilità di sfidare l'opposizione sulla necessità di rivedere gli stessi tre gradi di giudizio che un Paese moderno, avanzato, che vuole essere competitivo e che intende realmente dare alla sicurezza un valore di rango costituzionale, dovrebbe fare. Oggi ricorre l'anniversario della morte di Placido Rizzotto, un sindacalista, un socialista, che a Corleone, nell'immediato dopoguerra, si pose come un punto di riferimento nella lotta alla mafia; un punto di riferimento che voleva servire la sua piccola comunità, la sua terra (la Sicilia), il suo Paese, che aveva servito da partigiano a Nord, nella Resistenza, per costruire una classe dirigente capace di coniugare legalità e sviluppo.

Di fronte a questo scenario non c'è nessun grado di responsabilità capace di dire al Paese: usciremo dalla crisi migliori di prima perché ne stiamo curando i mali profondi, anche nel settore nel settore della giustizia. No, non c'è questa tensione. Non c'è una sfida lanciata all'opposizione per migliorare le condizioni del rapporto tra cittadino e giustizia. C'è ancora una volta l'idea arbitraria, discrezionale, rovinosa, di come il Presidente del Consiglio si rapporta con i suoi processi. Attenzione: non è vero che il dopo Berlusconi vedrà il nostro Paese rifiorire nella sua cultura giuridica, antica, istituzionale, perché i danni che si stanno causando vanno in profondità, scendono nei capillari del Paese fino a raggiungere le classi dirigenti. Queste ultime, tutte, si pensano all'interno di questo rapporto con il potere, che in Italia si costruisce con i privilegi e le impunità. È quello che sta avvenendo, signor Presidente, con tutti i casi che stanno deflagrando di fronte a noi e con tutti quelli che abbiamo potuto constatare

che hanno già subito delle condanne per fatti di mafia! Ecco che allora, di fronte a queste condizioni in molte Regioni

un provvedimento di questo tipo, il legittimo impedimento, un'arbitraria e insopportabile ricerca del Presidente del Consiglio di avere l'ennesima possibilità di aggirare i suoi processi, diventa uno scandalo e un punto vero di debolezza del sistema Paese. Noi lavoreremo per rimuoverlo con serietà e con progettualità e lo faremo oggi in quest'Aula così come lo faremo nel Paese, a partire dalle iniziative pubbliche che si stanno organizzando con la manifestazione che mi auguro possa diventare un grande evento democratico per la cultura politica del nostro Paese, nonché per la cultura politica dei moderati di questo Paese, che meritano una classe dirigente che li sappia guidare e che abbia in testa e nel cuore le sorti democratiche, lo sviluppo e la legalità dei nostri territori.

ma tutto il dibattito perché questa opposizione, dopo aver chiesto la presenza del Presidente del Consiglio,

che guardano soprattutto agli aspetti tecnici e giuridici di questo provvedimento. Io voglio sottolineare il fatto politico perché questo è un problema che ha radici politiche molto profonde e molto inquietanti.

in questo momento assistiamo ad una vicenda che ci porta a dire che in questo Paese le regole non hanno alcun valore; si sbaglia e si chiama sopruso quello che l'errore produce. La logica qual è? Qualsiasi accadimento, qualsiasi errore in questo Paese può essere sanato. Questa è la logica inaccettabile; logica che è stata recentemente fortemente contestata anche da autorevoli espressioni morali di questo Paese. Mentre il Paese vive il dramma della mortificazione dei diritti dei lavoratori, consuma il dramma di una crisi sociale che dovrebbe essere affrontata con maggiore determinazione, noi siamo impegnati da mesi, caro Ministro, su questa vicenda. Quanto tempo abbiamo perso sul processo breve, signor Ministro? Quante risorse di questo Parlamento sono state impegnate? Lo abbiamo affrontato per settimane e settimane; siamo intervenuti tutti in Commissione giustizia. Ad un certo punto vi rendete conto che il processo breve non serve e lo mettete da parte, in attesa di tempi migliori. Vi sembra un modo di rispettare il Parlamento o possiamo arguire facilmente che il Parlamento è completamente asservito alle esigenze del Capo del Governo? Una maggioranza allo sbando. Guardi, signor Ministro, avrei voluto che ieri fosse presente in Aula quando il suo collega Vito Vito ha annunciato la fiducia: c'era costernazione e disagio nei colleghi di maggioranza. Purtroppo il dramma è che il disagio dei nostri colleghi di maggioranza nel migliore dei casi si trasforma in mugugno clandestino, mai in parola e in azione. vero di questa nostra sfiducia, vale a dire l'impossibilità di un dialogo vero in quest'Aula. Vi siete spaventati dei nostri 1.200 emendamenti: cos'altro può fare un'opposizione

in segno di dispregio di ogni autonomia e di ogni autonoma prerogativa del Parlamento. Vedete, abbiamo usato spesso l'espressione «legge *ad personam*».

cui si parla apertamente di impedimento «continuativo e correlato allo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge». Sostanzialmente solo tre volte il Presidente del Consiglio dovrà dire che non può essere presente, e non perché è impedito ma perché è il Presidente del Consiglio. E noi non sappiamo quanto il Presidente del Consiglio sia oggettivamente e legittimamente impegnato. diciotto mesi. Se l'*iter* di riforma della Costituzione non andrà in porto sapete bene che fra diciotto mesi saremo di nuovo qua e vi inventerete un'altra cosa perché occorre assolutamente evitare che il *Premier* sia sottoposto, come tutti gli altri cittadini di questo Paese, alle leggi dello Stato.

Anch'egli è innocente, fin quando la legge non lo avrà definitivamente condannato. Che differenza c'è? Vi siete invece accaniti tutti ed

Siete stati forti con i deboli e deboli con i forti. In altri tempi il Paese avrebbe reagito, questa è la mia pena e la mia preoccupazione.

l'idea di fondo che guida la vostra azione di governo è che il consenso è superiore alle regole e allo Stato. Questa è un'idea eversiva *(Applausi dal Gruppo PD)*, questo è il fondamento e la legittimazione di ogni vostra azione!

verrebbe da citare anche in quest'Aula: «*Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra*?». Fino a quando? Ma la mia preoccupazione non è

è palesemente contrario ai princìpi generali dell'ordinamento e allo Stato di diritto. Oltre ai gravi aspetti già sottolineati da colleghi del mio Gruppo, il disegno di legge si applica infatti anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato e grado, alla data di entrata in vigore del disegno di legge. Si sancisce, pertanto, in violazione dei princìpi generali dell'ordinamento in materia di efficacia della legge nel tempo e dell'articolo 11 delle disposizioni preliminari del codice civile in particolare, l'applicazione retroattiva di norme procedurali ai processi iniziati sotto la vigenza di altre e diverse regole, laddove invece appartiene al secolare patrimonio del diritto il dato certo secondo cui la legge non dispone che per l'avvenire e non può avere pertanto effetto retroattivo, principio raccolto anche dai codici. La sospensione procedimentale prevista dal presente provvedimento è derogatoria rispetto al regime processuale comune, perché si applica solo a favore dei titolari di cariche governative, con riferimento ai processi instaurati nei loro confronti per imputazioni relative a tutti gli ipotizzabili reati extrafunzionali, cioè estranei alle attività inerenti alla carica ricoperta, commessi anche prima dell'assunzione della carica. La deroga si risolve come ricordato, da ultimo, nella sentenza della Corte costituzionale n. 262 del 2009 - in particolare in un'evidente disparità di trattamento delle cariche rispetto a tutti gli altri cittadini, che pure svolgono attività che la Costituzione considera parimenti impegnative e doverose, come quelle connesse a cariche o funzioni pubbliche, così come previsto dall'articolo 54 della Costituzione, o ancora più generalmente quelle che il cittadino ha il dovere di svolgere al fine di concorrere al progresso materiale o spirituale della società, così come previsto dall'articolo 4, secondo comma, della Costituzione. L'estendersi della sfera immunitaria dei soggetti detentori del potere politico con termini e modalità diversi rispetto ad altri cittadini rappresenta una lacerazione profonda del tessuto costituzionale repubblicano, una svolta culturale che tende a modificare la visione generale del sistema istituzionale complessivo, mettendo seriamente in discussione sia la forma di governo, e quindi i rapporti tra gli equilibri e i poteri, sia la forma di Stato, e quindi i rapporti tra il potere e i cittadini. La deroga al principio di non retroattività non vale per i cittadini comuni, ma solo per gli imputati che rivestono la carica di Ministro o Presidente del Consiglio dei ministri. La prerogativa si trasforma, nel provvedimento in oggetto, in privilegio e i privilegi sono ammissibili negli Stati costituzionali di diritto. Può, a tal proposito, evocarsi anche sotto il profilo della ragionevolezza la violazione dell'articolo 3 della Costituzione, signor Ministro; la discrezionale disponibilità della sospensione processuale, realizzata *de facto* mediante rinvio delle udienze, riconosciuta ai titolari delle cariche governative, si pone in contrasto con la tutela del *munus publicum*, attribuendo una discrezionalità meramente potestativa al soggetto beneficiario, anziché prevedere quei filtri aventi carattere di terzietà e quelle valutazioni delle peculiarità dei casi concreti che solo, secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2004, potrebbero costituire adeguato rimedio rispetto all'automatismo generalizzato del beneficio, quanto al *vulnus* del diritto di azione. Rispetto ai provvedimenti concernenti la materia giustizia, esaminati durante la legislatura in corso, di veramente innovativo nel presente disegno di legge sembra esservi proprio il citato articolo 2, laddove si legge che la disposizione in esame pretenderebbe di costituire un ponte rispetto all'approvazione con legge costituzionale di una norma scudo costituzionalizzata, appunto. Si è di fronte ad una norma a scadenza, che peraltro viene illogicamente applicata ai reati comuni ed esclusa per i reati funzionali e per i quali l'impedimento, configurato all'articolo 1, commi 1 e 2, non sarebbe invocabile. Lo scudo verso cui il disegno di legge in esame getta un ponte potrebbe essere rappresentato dal contenuto cosiddetto lodo Alfano, ripresentato magari in forma di legge costituzionale, oppure dal ripristino *sic et simpliciter* dell'immunità parlamentare. Tuttavia siffatto annuncio, lungi dal rappresentare una legittimazione costituzionale della legge, ne confessa il contrasto con la Carta costituzionale, così come lo sblocco finale possa essere rappresentato solo e soltanto da una legge costituzionale, approvato con le modalità di cui all'articolo 138 della Costituzione. Detta premessa legislativa costituisce, quindi, un'attestazione esplicita della incostituzionalità palese del provvedimento in oggetto. Si tratta non di una legittima disciplina del processo rimessa al legislatore ordinario, ma di una forma di deroga al normale esercizio della funzione giurisdizionale, che solo il legislatore costituzionale potrebbe eventualmente stabilire. L'impedimento legittimo è, infatti, per sua natura, qualcosa di puntuale e concretamente localizzato nel tempo: una presunzione *ex lege* assoluta di impedimento "continuativo" per un lungo periodo di tempo equivarrebbe ad una norma di *status* derogatoria, Peraltro il provvedimento contraddice se stesso nella parte in cui si riconosce che servirebbe una legge costituzionale ma poi fa rinvio all'articolo 2 che lo nega. Si tratta di una violazione palese del contenuto delle sentenze della Corte costituzionale sul lodo Alfano e sul lodo Schifani, signor Ministro: una violazione effettuata con una nuova legge incostituzionale. *(Applausi *(PD)*. Signor Presidente, devo confessare che faccio questo intervento con un sentimento di umiliazione democratica.

è la prova di un'arroganza senza fondamento, un'offesa alle prerogative del Parlamento. Ci sono solo due articoli.

discutere di questi emendamenti nel merito, giudicarli ed approvarli? Non c'era alcun motivo tecnico che impedisse di fare questo lavoro. Mi consenta, che anche lei, signor Presidente, mi ha deluso, perché non ha difeso le prerogative del Parlamento. Certo, non ha alcuno strumento regolamentare per obbligare il Presidente del Consiglio, ma ha la capacità persuasiva della seconda carica dello Stato. Prima ci ha detto che i Ministri erano presenti: i Ministri sono stati presenti solo quando c'era bisogno di votare e resta qui solo un Ministro. Nei giorni scorsi sulla stampa regionale è apparso un intervento del professor Mario Bertolissi, un insigne costituzionalista, allievo prediletto del professor Paladin, già Ministro e già Presidente della Corte. Diremmo un uomo moderato, una persona che collabora con il vostro Governo, che è stata consulente della Presidenza Galan della Regione Veneto e che è stata proposta dal centrodestra come possibile candidato al Comune di Padova. Commentando il decreto sulle liste il professor Bertolissi ha scritto: «Dichiaro il mio disprezzo per chi fa strame delle regole fondamentali della convivenza. Distruggere il senso della legalità mi sembra rappresenti il delitto istituzionale più efferato, perché alimenta la corruzione delle coscienze». Perché un uomo moderato come il professor Bertolissi usa toni così forti e dà voce anche a tanti vostri elettori del passato? Perché il troppo è troppo, signor Presidente. Il tutto si inserisce nella torsione di un'agenda politica che porta a negare con sovrana indifferenza perfino l'esistenza di una grave crisi Si minimizza, si nega. Il Paese, nei suoi lavoratori, nei suoi imprenditori, nei suoi professionisti, sta soffrendo questa crisi e dal Governo non riceve non dico la soluzione, ma neppure il riconoscimento che sta soffrendo e sta lavorando per portar fuori il Paese dalla crisi. Il troppo è troppo. Ieri, appunto, le norme sulle liste. L'altro ieri avete consentito che circuiti criminali e paranazisti manipolassero le elezioni e portassero qui dei parlamentari. Non avete difeso l'onorabilità del Parlamento; avete fatto finta di non vedere e di non sentire. *(Applausi dal Gruppo è dovuta intervenire perché voi non siete stati capaci di difendere l'onorabilità della politica. Il troppo è troppo. Vi è lo scandalo della Protezione civile, i cui confini, certo, saranno accertati dalla magistratura, ma che svelano comunque pesanti complicità, mancate vigilanze, che hanno consentito che pezzi di poteri pubblici costituissero una organizzazione criminale. Perché di questo si tratta: una organizzazione criminale nata nell'ombra delle istituzioni. E badi, signor Presidente: il Governo non ha ancora pronunciato una parola per scusarsi nei confronti delle centinaia di migliaia di volontari che hanno fatto grande la Protezione civile e che sono offesi dal lievitare all'interno di quella struttura del malaffare. Le uniche parole che ha usato il Presidente del Consiglio sono state per offendere i magistrati che hanno dimostrato l'esistenza di questo circuito criminale. Solo la determinazione dell'opposizione ha consentito che voi non poteste completare un disegno finalizzato a stendere una rete di protezione assoluta attorno a questo circolo criminale. Allora il troppo è troppo e il troppo è troppo anche con questo provvedimento. Un altro grande pasticcio. Siete riusciti a far diventare di parte una questione che è una grande questione della democrazia: la possibile esistenza di garanzie particolari per le diverse funzioni, per i diversi poteri dello Stato che solo la Costituzione può regolamentare come eccezione al principio di eguaglianza di fronte alla legge. Non c'è un legittimo impedimento, non può esserci un legittimo impedimento basato sulla illegalità. Non può esserci nulla di più illegittimo della pretesa di un'immunità individuale al di fuori della Costituzione. Vede, signor Presidente, nei giorni scorsi ero col senatore Bosone a Pavia per una manifestazione politica. Abbiamo visitato la bella chiesa di San Pietro in Ciel d'Oro a Pavia, che ospita le spoglie mortali di Severino Boezio, il grande umanista cristiano assassinato dal potere costituito nel V secolo perché voleva difendere la libertà, aveva questa presunzione di difendere la libertà. In una delle sue opere scritte in carcere mentre attendeva la pena di morte lascia questa notazione: «Quei re che vedi assisi in alto trono, di porpora splendenti, d'arme cinti paurose. Se togli a quei superbi vani pregi il velo vedrai che nel profondo sono avvinti da assai strette catene». Noi pensiamo che lo splendore della porpora di questo consenso consenso così forte nel Paese, di questo potere di ricatto le armi paurose stiano venendo meno e i cittadini si accorgono che le strette catene di un'agenda tutta distorta sugli interessi personali di una persona sono inadatte a consentire la guida di questo Paese. Siamo qui per difendere il valore di quella patria comune del diritto che è la nostra Costituzione e ci auguriamo che le prossime elezioni costituiscano per tutti i cittadini lo strumento per difendere insieme questo valore costituzionale. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghe senatrici e colleghi senatori, credo che dobbiamo interrogarci, come ha fatto poco fa il collega Gerardo d'Ambrosio, sul perché il Parlamento è bloccato dai problemi giudiziari del Presidente del Consiglio che non può affrontare le gravi questioni relative alla crisi che sta investendo Lo diceva anche la nostra presidente Anna Finocchiaro questa mattina. Per chi avesse dei dubbi si legga le rilevazioni di opinioni Ipsos de «Il Sole 24 Ore» sulle Regioni. In questo momento i nostri cittadini sono letteralmente angosciati dai problemi di lavoro, della crisi economica. Il vostro Governo, signori che state lì seduti su quei banchi, è quello che nei Paesi occidentali ha fatto di meno nonostante le sollecitazioni che vi abbiamo rivolto, e noi siamo qui fermi da mesi per affrontare esclusivamente provvedimenti legati alle vicende giudiziarie del Presidente del Consiglio. È già stato fatto l'elenco dal 2001: le rogatorie internazionali, il falso in bilancio, la riduzione dei termini della prescrizione con la legge Cirielli, il lodo Schifani, poi lodo Alfano, giudicati incostituzionali, per la protezione la protezione dai processi delle alte cariche dello Stato durante lo svolgimento delle proprie funzioni. Ma perché? Perché tutto questo nonostante più volte questi provvedimenti siano poi caduti La mia risposta è che voi siete prigionieri della vostra stessa ideologia, cioè dell'idea secondo la quale è sufficiente avere il consenso elettorale per essere liberati da qualunque regola e da qualunque controllo. È un'idea populista, che dall'interno della vostra stessa maggioranza viene finalmente contestata, contraria ai principi fondamentali dello Stato di diritto e della cultura liberale, quelli ai quali è ispirata la nostra Costituzione e che prevedono che ad un potere esecutivo corrisponda un potere legislativo in grado di indirizzarlo e controllarlo, e un potere giudiziario autonomo nell'esercizio delle proprie funzioni. È ciò che vi ha portato anche al decreto salva liste: un provvedimento pasticciato, costruito con l'esclusiva volontà di risolvere il problema che in quel momento avevate senza badare al fatto che calpestavate la legge e la Costituzione, come giustamente vi è stato ricordato dai tribunali che si sono pronunciati in questi giorni sull'ammissione delle liste del PdL provinciale di Roma. Siamo qui oggi perché la Corte costituzionale nell'ottobre scorso ha dichiarato l'incostituzionalità del lodo Alfano. Da quel momento, il processo breve e con il legittimo impedimento, si è voluto porre rimedio sempre ed esclusivamente per affrontare i problemi giudiziari del Presidente del Consiglio. E lo si è fatto, ancora una volta, con strumenti che violano la legge e la Costituzione. Qui mi riferisco alla relazione di minoranza del collega Casson il quale, molto puntualmente, ricorda come vi sia già un articolo del codice di procedura penale, il 420-*ter*, che regolamenta la materia la materia del legittimo impedimento. In questa materia è necessario mantenere l'equilibrio tra l'esercizio della funzione giurisdizionale - tra l'altro siete voi quelli che volete fare, come noi, peraltro, ma sul serio, i processi brevi e in questo caso invece li allungate indefinitamente - e l'interesse l'interesse legittimo di chi ha funzioni pubbliche a che vi sia una continuità nel loro svolgimento. Voi alterate con il legittimo impedimento, così come ce l'avete qui presentato, questo equilibrio, introducendo una prerogativa assoluta per i membri del Governo. Ciò viola il principio di eguaglianza previsto dalla Costituzione e non può che incorrere di nuovo nella sanzione di incostituzionalità della Corte che sarà sicuramente interpellata. Infine, voglio soffermarmi anch'io, come hanno fatto altri colleghi, sull'abnormità dell'articolo 2 che stabilisce - è un'innovazione assoluta nel nostro ordinamento - il concetto di legge ponte, legge ponte, giustamente definito come una confessione di incostituzionalità da parte della maggioranza che lo propone su questo provvedimento. Ma l'abnormità arriva al punto di definire i caratteri che dovrà avere la modifica costituzionale, in quanto si parla si parla di una disciplina organica delle prerogative del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri. Bene, il collega D'Ambrosio ha avanzato nel corso delle scorse settimane, e ricordato oggi in quest'Aula, una soluzione possibile non del problema del Presidente del Consiglio ma di quello del rapporto tra politica e magistratura, come diceva giustamente anche il senatore Giaretta, utilizzando quelle prerogative che solo la Costituzione può prevedere

percorsa: prevedere costituzionalmente, intervenendo sul tema delle immunità, la possibilità per gli eletti in Parlamento e per i membri del Governo di sospendere i propri processi per una sola legislatura, nell'ultimo anno di essa di avere una corsia riservata per affrontare il giudizio, con l'obbligo di non ricandidabilità qualora non venissero risolti i propri problemi con la giustizia. Questa, che potrebbe essere una soluzione, voi non

I colleghi dell'Italia dei Valori, avendo convocato tutta la stampa, che altro non fa che indicare in loro l'unica opposizione a questo pessimo Governo fascista di Silvio Berlusconi, in silenzio, quindi senza violazione (o ancora siamo di fronte ad una interpretazione che lei, Presidente, mi pare, abbia dato, dicendo che non vi è stata violazione degli articoli 66, 67 e 68, perché non ha richiamato all'ordine nessuno), come hanno fatto negli ultimi due anni e mezzo tutte le volte che noi, radicali, abbiamo denunciato la violazione quotidiana e sistematica della nostra Costituzione, si sono messi a sedere nell'emiciclo. Ciò sta turbando i lavori fino ad un certo punto perché, non essendoci nessuno in Aula, è chiaro che non s'impedisce a molti di tornare al proprio posto per ascoltare questo dibattito. Spero che decidano di rimanere ed occupare l'Aula nella pausa pranzo, almeno fino alle ore 17, quando il gioco, in effetti, si farà duro e dovranno votare no alla fiducia di questo Governo fascista di Silvio Berlusconi, che calpesta quotidianamente la Costituzione. Spero anche che se lo ricordino dopo le ore 18, quando correranno a prendere l'aereo per tornare a casa. La lotta per salvare la Costituzione dall'attentato, che non va avanti da un anno e mezzo, ma da almeno tre decenni, va portata avanti quotidianamente, non con le pagliacciate *una tantum* a reti unificate (e qui ci sono sicuramente tutte le televisioni a vedervi): va portata avanti militantemente, anche con l'uso della non violenza, salvo poi aggregarsi al carro dei «vincitori», a coloro cioè che cercano di attivare quel minimo di legalità ancora consentito in questo Paese, e di far emergere la sistematica violazione dei diritti civili e politici degli italiani. Questa legislatura si è aperta con un caso

adesso egli deve rispondere di fronte alla giustizia. Questa sistematica violazione dello Stato di diritto è continuata, aggravandosi di giorno in giorno.

trasferendosi in uno dei tre forni che li caratterizza: nel forno di maggioranza, quello che sostiene il Governo di Silvio Berlusconi, grande nemico della Costituzione. Si devono assumere la responsabilità di aver partecipato a che cosa?

Cari colleghi dell'Italia dei Valori (che più di altri sono attenti al rispetto della Costituzione in piazza e negli emicicli, ma magari meno nell'attività politica parlamentare, in quanto partito),

dell'UDC e anche senza la nostra opposizione, sarebbe stato comunque portato a casa. In Italia occorre un'amnistia nei confronti della violazione dello Stato di diritto e delle omissioni gravissime di questo Governo, buon ultimo, e di quelli degli ultimi trent'anni contro le violazioni dei diritti individuali. Per questo voteremo no alla fiducia: ma credo che il no vada anche contro gli atteggiamenti cosmetici di buona parte della minoranza.

Sempre in questo testo si fa riferimento - e potrei concludere così data l'autorevolezza del professor Cordero - alla "burla degli impedimenti" e c'è uno specifico capitoletto dedicato al tema di cui stiamo discutendo.

perché il TG1 è scandalosamente assente dalla vicenda politica italiana; parla d'altro, di cellulari tuttofare, di notizie pseudorosa, ma non della drammatica vicenda che qui stiamo vivendo. Così anche suona sospetta oggi più che mai l'eliminazione da parte di una dura ed ispida maggioranza autoritaria del consiglio d'amministrazione della RAI di quelle rubriche di informazione che forse avrebbero potuto ospitare con la *par condicio* va da sé - autorevoli o meno autorevoli esponenti del mondo politico e del mondo associativo della società per comprendere e far comprendere, dibattere ed approfondire un argomento che suona curioso persino a chi di queste cose ha cercato di occuparsi. Che cosa è esattamente questo legittimo impedimento? Ora, scorrendo questo breve testo normativo (certo è piuttosto veloce questo articolato e certamente ha un'interpretazione più semplice di altre più complicate vicende legislative), leggendo questo testo balza immediatamente agli occhi una contraddizione persino plateale tra

che assomiglia sempre più a quei tratti che Antonio Gramsci ben chiariva con sintesi efficace con l'espressione "sovversivismo dall'alto". Da una parte, quindi, c'è un vantaggio inaudito anche questa volta *ad personam*, a favore di varie persone. Mi riferisco a quello contemplato in un'ennesima forma di viatico del potere

Quindi, in un certo senso in questi due articoli si contiene il testo e il suo contro testo, quasi come in una celebrazione situazionista o futurista in cui al testo iniziale si accompagna l'eliminazione di quel testo stesso.

con motivazioni totalmente improbabili che potevano valere per questo come per la botanica e per qualche altro argomento, il ministro Vito ha evocato la fiducia mi sono chiesto perché mai si è scelta l'urgenza della fiducia di fronte a una proposta di legge piuttosto succinta che poteva essere regolata in qualche ora di dibattito. Mi avvio a concludere Presidente, Ministro, colleghe e colleghi, e spero che il tono della voce, pur contenuto, tradisca - vorrei che fosse così - un'amarezza come parte di questo bel Paese. In verità questa è, infatti, una delle tante iniziative che nella società mediatica e post-mediatica - qualcuno meglio di me ha indagato questo processo - vogliono entrare non tanto e solo nell'ordine politico e istituzionale delle questioni - se così fosse sarebbero più circoscritte nel loro danno - ma in quella complessa e articolata categoria che è l'ordine simbolico: per dare l'idea che si può fare tutto, che non c'è alcun remora. Così com'è stato anche per il decreto cosiddetto "salvaliste", che ha avuto un esito non così felice, si deve un esito non così felice, si deve dare simbolicamente un messaggio alla società italiana tutta e anche a coloro che non sono ancora convinti e che sono un po' eretici rispetto al potere che si può fare qualsiasi cosa e che non c'è regola che tenga e che per chi è dentro quel fortilizio tutto il resto è secondario.

ero quasi improvvisato utopista e dicevo: in fondo forse sarà perché c'è di mezzo la televisione, il resto andrà meglio. Invece non è così e mi sto accorgendo che quelle vicende di allora, dal decreto Craxi in poi, insomma tutto quello che ha costituito la premessa per ciò di cui viviamo oggi le conseguenze, non era altro che la prefigurazione, la premonizione di una fondamentale "nuova normalità"; la normalità del male, come tante volte e bene scrittori rilevanti - ne cito una, Hannah Arendt, che sta cuore a tutti noi - hanno scritto. Non dobbiamo adagiarci, non possiamo arrenderci e noi dall'opposizione non ci arrenderemo. Potrà anche passare con la fiducia questa legge, ma sarà presto stracciata dalla realtà delle cose.

Lo dimostra, tra l'altro, il comma 4 dell'articolo 1, su cui incentrerò il mio intervento, che prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri (attribuendo quindi tale delicata funzione alla struttura organizzativa di supporto del Presidente-imputato) attesta, di fatto con effetto vincolante per il giudice, che l'impedimento risulta essere "continuativo" in relazione alle funzioni svolte, senza indicare il criterio o il parametro con cui commisurare questa discrezionale attestazione, e quindi rendendo l'applicazione della legge arbitraria ed imprevedibile. Si presume, per quanto non specificato, che l'attestazione della Presidenza possa valere sia per il Presidente del Consiglio che per i Ministri. Siamo davanti, quindi, ad una autocertificazione amministrativa - o meglio, governativa - assoluta, che consegna in mano all'imputato, Ministro o Capo del Governo, il calendario delle udienze, ben al di là di quei fatti imprevedibili di assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito o forza maggiore che renderebbero legittimo l'impedimento. Sempre con il comma 4 si introduce nella legge anche un ulteriore elemento. L'imputato potrebbe prevedere e anzi contribuire a determinare l'impedimento e quindi ci troveremmo da una parte davanti a qualcosa di molto lontano dalla natura dell'impedimento conosciuto dal codice di rito, inteso come fatto al cui verificarsi ne conseguano effetti impeditivi non prevenibili e non previsti dall'imputato, e dall'altro si sottrae al giudice la possibilità di verificare, giorno per giorno, la sussistenza e la costanza delle ragioni impeditive. Analoga valutazione può esser fatta per le attività "consequenziali" che, ai sensi dell'articolo 1, costituirebbero altro legittimo impedimento a comparire in udienza. Quindi, mentre a qualsiasi cittadino imputato che deve comparire davanti al giudice viene richiesto di circostanziare l'eventuale impedimento, il Presidente del Consiglio, invocando genericamente le sue attribuzioni, potrà programmare con anticipo i suoi impedimenti e richiedere ed ottenere di non presentarsi al cospetto dei giudici e dunque di non farsi processare. Il comma 4, inoltre, fissa un termine semestrale massimo di rinvio, astrattamente individuato e non motivato da alcun elemento fattuale, secondo una logica che non sembra però sposarsi, almeno dal punto di vista della coerenza, neppure con lo stesso concetto di continuatività introdotto dal comma 4 medesimo. Infatti, se si volesse ammettere l'esistenza di situazioni impeditive continue - ammesso che si possa superare l'obiezione della oggettiva prevedibilità di tali eventi non si vede come tale continuatività sia ragionevolmente riconducibile al termine dato (sei mesi) peraltro reiterabile (fino a tre volte) quasi a configurare un impedimento semipermanente, la cui permanenza viene però constatata non dal giudice bensì da chi ne beneficia. Quindi con il comma 4 si stabilisce, per legge, che ci sarà in futuro e per un dato periodo di tempo un impedimento a comparire, quando invece il fatto impeditivo impeditivo dovrebbe verificarsi prima delle sue conseguenze (l'impedimento a comparire) o, quanto meno, con modalità non controllabili dall'imputato. Un termine di sei mesi - per non parlare dei diciotto mesi di validità complessiva della legge invece di per sé e con assoluta chiarezza che vi è, in questo lasso di tempo, ampia possibilità per l'imputato di organizzare adeguatamente i propri impegni ed assicurare così la presenza alle udienze che lo riguardano. Il comma 4, laddove fa riferimento a futuri impedimenti che non sono conoscibili e valutabili dal giudice al momento in cui essi vengono attestati dalla Presidenza del Consiglio, costituisce un fattore ulteriore che, insieme alla misteriosa correlazione dell'impedimento alle funzioni, contribuisce a ricondurre l'impedimento esclusivamente alla carica e non a specifiche attribuzioni o all'esercizio di precise funzioni inerenti la carica medesima. Anche la terminologia utilizzata contribuisce a rendere il comma 4 in questione particolarmente oscuro e contraddittorio: l'impedimento continuativo, infatti, secondo questo comma, deve essere anche «correlato all'esercizio delle funzioni» mentre come secondo il comma 1 - deve essere coessenziale alle funzioni di governo. Nella Costituzione, agli articoli 68, 90 e 96, l'immunità trova il fondamento ed il limite nell'esercizio della funzione. La Costituzione porta a ritenere strumentale ogni tipo di immunità riferita alla funzione esercitata. In base all'articolo 96 della Costituzione, l'autorizzazione a procedere può essere negata solo nei casi ivi previsti. Il nostro ordinamento costituzionale non prevede alcuna ipotesi di immunità personale, che si tradurrebbe in privilegio; privilegio che invece voi state ratificando per il Presidente del Consiglio e per i Ministri, stravolgendo ancora una volta i princìpi della nostra Carta fondamentale e ignorando i ripetuti richiami della Corte costituzionale, rimasta ormai quasi l'unico efficace baluardo della democrazia. Per questo, signor Presidente, noi dell'Italia dei Valori stiamo oggi facendo un *sit-in* pacifico, e non violento - come qualcuno ha voluto insinuare

quei momenti della vita di una comunità, di uno Stato, nei quali bisognava assolutamente fare il punto della situazione. Bisognava cioè fermarsi a pensare, a riflettere per cercare di far emergere dalla riflessione una valutazione oggettiva sulla realtà che

vorrei citare il vecchio catechismo che dava una precisa definizione del peccato mortale. Questa maggioranza, con piena avvertenza e deliberato consenso, stia facendo strame della nostra Costituzione, stia, cioè, saccheggiando un impianto giuridico che ha costituito - bisogna ricordarlo - il primo vero effettivo momento di incontro delle sensibilità degli italiani. Potremmo definirlo il primo vero compromesso storico. Che cosa sta facendo, tanto per restare alla materia? Si sta impegnando a costruire - possiamo chiamarla in tal modo - una «immunità a prescindere» per il Capo del Governo. Si sta arzigogolando in maniera molto efficace per ciò che riguarda il risultato, spudoratamente, superando ogni forma di decenza, pur di costruire intorno a quest'uomo una armatura, una sorta di scafandro grazie al quale poter attraversare impavido un percorso che altrimenti gli sarebbe stato precluso. Lo si vuole porre di fatto, signor Presidente, al di sopra di tutti e forse anche al di sopra del bene e del male. Signor Presidente, signor ministro Alfano, ho sentito anche lei in più occasioni, così come alcuni suoi colleghi, parlare in questi termini: - eravate voi che parlavate - «siamo il partito dell'amore, i figli della luce,

da pormi francamente qualche problema riguardo alla vostra effettiva capacità di discernimento, almeno per quanto mi riguarda - ma per fortuna so di non essere solo - vorrei dirvi che queste fesserie convincono soltanto voi.

Ma davvero, davvero, pensate che siamo così scemi da ritenere soltanto per un attimo che siate in grado di metterci in difficoltà, in crisi esistenziale perché voi siete il partito dell'amore, i figli della luce, gli apostoli del bene e noi esattamente il contrario? Dunque, senza timidezza, signor Ministro, affrontiamo anche questo altro passaggio di tempo e lo facciamo a testa alta, convinti che, auspicabilmente, nella vita di una persona, certamente in un paio di generazioni, ci sono momenti diversi che si realizzano. Se guardassimo, signor Ministro della giustizia, e sodali, che danno anche le spalle in maniera maleducata,

Cosa sono, in fondo, se non delle persone ingenue quelle che continuano a chiedere il numero legale, che ancora non si sono convinte che non è vero che la sostanza prevale sulla forma, perché la forma in uno Stato di diritto è sostanza; che non è vero che esiste un processo ineluttabile che i liberisti ladroni chiamano liberismo o globalizzazione e che gli innovatori chiamano segni dei tempi in ragione dei quali bisogna cambiare le regole del gioco e così, come state facendo in questi giorni, anche truffare il Paese. Che pena sentire certi rappresentanti del Partito arrampicarsi sugli specchi in maniera così patetica e oltraggiosa da permettersi di dire che è colpa della sinistra se stanno succedendo queste cose; che è colpa della sinistra se ci si sbaglia nel preparare le liste; che è colpa della sinistra, o dei comunisti, se si è talmente incapaci nella predisposizione di semplici incombenze di carattere elettorale da volersi proporre per la guida del Paese. Ecco, questo è uno di quei passaggi di tempo, signor Presidente, nel quale è bene ricordare che noi abbiamo uno sguardo rivolto oltre il presente e sappiamo - sempre per citare lo stesso poeta - che passerà anche questa stazione. Purtroppo passerà facendo male, ma passerà anche questa stazione e verrà il momento del *redde rationem*. Allora, anche quei tromboni che come me, magari in un'Aula distratta, parlano per lamentare i dolori per una Costituzione afflitta, forse potranno dire che il loro passaggio il loro passaggio di tempo non è stato inutile. Attenzione, perché potete pensare di ingannarci adesso, ma il popolo non lo state ingannando.

Senatore Caliendo, la invito a prendere posto nei banchi del Governo, per cortesia.

in questa fase del dibattito sulla questione di fiducia posta; ci sono senatori che giustamente, invece che stare a sedere nei loro scranni, stanno seduti per terra, voltando tranquillamente le spalle al Presidente del Senato, che non si accorge di nulla o, meglio, dà incarico ai senatori Questori di trattare non si sa che cosa. Cosa dovrebbe fare un Questore? Deve forse chiedere loro se hanno bisogno di una Coca-Cola, o di un panino, come va di moda in questi giorni, o qual è il problema che possono avere in questo momento? È evidentemente un problema politico, ma non si può intervenire sull'ordine dei lavori. Lei ha appena richiamato il senatore Longo, Presidente, che evidentemente ha avuto anche lui questa mala pensata di essere in Senato; non si può più intervenire sull'ordine dei lavori ma soltanto in merito - anche questo abbastanza

perché non si attagliano bene a quel caso specifico che si intendeva risolvere. D'altra parte, quando si fanno le cose così mal fatte e dettate dalla fretta per un'esigenza particolare e peculiare, poi accade anche che questi

Non sarebbe questo certo il problema. Se invece il provvedimento è fatto solo per una persona, anche se in questo momento quella persona è il Presidente del Consiglio,

troviamo, invece, ad inseguire l'emergenza del Berlusconi di turno, in uno scontro che non avrà mai fine, in un gioco delle parti tra la magistratura ed il Presidente del Consiglio, i quali non possono fare altro che tirarsi calci negli stinchi ogni volta che ne hanno l'opportunità, tradendo completamente lo spirito della Costituzione e affondando del tutto lo Stato di diritto. Quindi, mi auguro davvero che il ministro Alfano, (se tornerà), ci ragguagli sulle intenzioni della comunità internazionale nei nostri confronti*.

Sì, lo farò. Prendo atto e subisco questa imposizione, che viene fatta da persone che non rispettano il diritto degli altri senatori a svolgere il proprio intervento in una condizione di normalità. Voi non rispettate il mio intervento!

clima ci si vuole sottrarre a un puro argomentare propagandistico. Tuttavia c'è una domanda dalla quale voglio partire: quando i cittadini, o gran parte di essi, vedono nella politica un ostacolo e non una risorsa rispetto ai loro problemi, si sbagliano? Sono in preda al qualunquismo o parlano di una cosa reale? Noi - non voi - cosa stiamo facendo di fronte a questa situazione?

Questa legge ci parla di un Presidente del Consiglio e di un Governo che lui guida che hanno ormai rinunciato a qualsiasi ambizione di trasformazione, dominati dai *Premier*. Altro che vittima di un complotto! Ci parla di una persona vittima delle proprie ossessioni. So quanto Berlusconi sia ricco e potente, naturalmente non ignoro questo; ma se osservo la situazione, mi pare di vedere invece un poveruomo che non sa più che pesci prendere, che non sa più dove andare, che si agita in modo scomposto, provocando danni che poi sarà molto difficile riparare. È come coloro che di fronte ad una storia esaurita non sanno come mettere la parola fine; come quei tanti - è capitato anche a me - che quando prendono la parola e fanno un discorso non sanno come concluderlo e vanno avanti in questo modo. Siamo in questa situazione. Mi pare che che la fiducia confermi questo fatto, cioè che prevalga in voi, coinvolgendo in questo tutti, l'attesa inerte di una fine i cui segnali sono sempre più evidenti. Anche la vicenda delle liste - lasciatemene parlare - è esemplare da questo punto di vista. È ovvio che dietro la questione delle liste, che contribuisce così tanto ad inasprire il confronto politico in questo momento, vi è una questione di regole; ma guardate che il problema principale non è una questione di regole, bensì di sostanza. Provate per un attimo a cambiare il posto che ciascuno di noi occupa e a guardare da un altro punto di vista questa realtà; provate a immaginare che non sia stato il PdL a sbagliare la presentazione delle liste a Roma, ma che sia stato il Partito Democratico

trova la gran parte dei problemi che stiamo affrontando. Se lo avessimo fatto noi per voi, o voi per noi, è evidente che il provvedimento sarebbe stato del tutto costituzionale, perché la Costituzione non è solo un insieme di regole, ma è anche una spinta verso l'equità, la giustizia e l'imparzialità nell'uso del potere. È tutto questo che oggi è in discussione. Cercare una soluzione politica avrebbe avuto un senso, perché significava affrontare questo problema. riconoscere un errore non era semplicemente la pretesa di incassare rapidamente qualcosa da spendere sul mercato elettorale nelle prossime settimane, ma era la premessa per affrontare una discussione politica seria, di cui non abbiamo bisogno noi o voi, ma di cui ha bisogno il Paese in questa crisi politica. Quello che è incostituzionale non è mettere mano alle regole quando questo è necessario: quello che è incostituzionale nella sostanza è farlo solo per se stessi, è eludere un confronto che su questo rappresenti un punto d'equilibrio per i cittadini. Questa è a mio parere la questione essenziale. Naturalmente, quando di fronte a tale questione c'è qualcuno che parla di *impeachment* del Presidente della Repubblica penso che si tratti solo di una mascalzonata politica. Gruppo PD)*. Oggi su questo episodio, se non siamo ciechi, possiamo leggere una sintesi della situazione politica italiana e dell'*impasse*, della paralisi nella quale tutti siamo. Con il voto di fiducia di oggi e con gli atti politici che state compiendo in questi giorni voi mettete in evidenza quello che, io dico purtroppo, siete diventati: un ostacolo per un Paese che ha bisogno di cambiare*.

tutti i colleghi dell'Assemblea che il Gruppo dell'Italia dei Valori sta seguendo con molta attenzione lo svolgimento e la prosecuzione di questo importantissimo dibattito, dibattito, che coinvolge in modo particolare tutti gli italiani. Voglio altresì ringraziare il senatore Perduca per gli utili, importanti, preziosi consigli di democrazia e di impegno civile che, provenendo da chi ha avuto come segretario nazionale di partito per diversi anni l'onorevole Capezzone, che è uno dei massimi esperti della democrazia nel nostro Paese, rappresentano

e Berlusconi, il provvedimento sul legittimo impedimento era il prezzo giusto da pagare. è la valutazione del disegno di legge che dà la terza carica dello Stato; questo è il ruolo del Parlamento a cui questa maggioranza di centrodestra ci sta abituando ormai da troppo tempo: non a fare leggi nell'interesse generale o per il bene comune, ma leggi che abbiano il prezzo giusto. A queste straordinarie scolaresche che vengono qui ad assistere al lavoro del Parlamento noi stiamo insegnando che questa maggioranza di centrodestra sta cambiando lo Stato di diritto in uno Stato di mercato del diritto: uno Stato di mercato del diritto dove chi ha più soldi, più potere, più forza, più arroganza può acquistare i diritti di cui godere, le funzioni e le attribuzioni cui assolvere e le prerogative di cui usufruire. Questo è quello a cui si sta riducendo il nostro Paese: lo Stato del mercato del diritto. Vede, signor Presidente, vogliamo accogliere il suo monito che, provenendo dalla seconda carica dello Stato, richiede anch'esso molta attenzione. Lei dice che, in fondo, in democrazia ciò che conta è la sostanza e non la forma, anche se poi i Padri costituenti ci hanno insegnato che la forma come rispetto delle regole e delle procedure è essenza stessa della democrazia. E dispiace che alcuni colleghi si accorgano di come la forma

restiamo alla sostanza delle cose. Signor Presidente, questo disegno di legge non ha i piedi per camminare, e lo sa tutta l'Aula. Ma voi pensate che all'interno della maggioranza, dove vi sono importanti costituzionalisti, non si sappia che questo disegno di legge

E se andiamo sui singoli commi, il comma 1 dell'articolo 1 avrà bisogno - e lo sapete tutti - di un decreto interpretativo. La cosa ci preoccupa, perché l'esperienza e la competenza di questo Governo sui decreti interpretativi la stanno sperimentando tutti gli italiani. È pacifico, che un Presidente del Consiglio abbia un legittimo impedimento per le funzioni che gli vengono attribuite da leggi e da regolamenti, ma diventa di difficile interpretazione quando si dice che questo legittimo impedimento ci sia anche per attività che sono coessenziali alla funzione di governo. È sulla coessenzialità che cade tutto il problema. Vedete, giorni fa il Capo del Governo ha dichiarato al TG1 e al TG2 che sarà presto in visita in Campania insieme al maestro Apicella in quanto dovrà, dopo avere composto una canzone, cantarla alle popolazioni della Campania. Vi chiederete: ma questa è una funzione coessenziale? Per me sì, perché è da ricondurre nella fattispecie della promozione da parte del Capo del Governo della cultura, dell'arte, della musica. per qualche giudice talebano infiltrato all'interno della Costituzione può essere considerata una funzione coessenziale? Qui è allora il problema. Sul comma 2, vi è la schizofrenia del considerare 22 Ministri importanti per l'attività del Governo: penso al ministro Gelmini, che sta tagliando scuola, università, ricerca. Ai Ministri va garantita una immunità permanente per diciotto ai poveri Sottosegretari non viene garantita nessuna immunità. L'apoteosi poi si raggiunge con l'articolo 2, dove, rispetto alla democrazia americana, *(IdV)*. Mi avvio alla conclusione. Rispetto alla Costituzione americana, che prevede l'attenzione verso la felicità di tutti i cittadini, noi con l'articolo 2 prevediamo il diritto alla serenità del Capo del Governo e di 22 Ministri. Il diritto alla serenità: anche questo sarà un intoppo di fronte alla Corte costituzionale, perché non vi è giurisprudenza che chiarisca cosa è questa serenità. I vocabolari italiani dicono che la serenità è uno stato d'animo di tranquillità, lontano da preoccupazioni, da noia e da rimorsi.

sulle noie del Capo del Governo non c'è bisogno che gli diamo consigli perché sa provvedere autonomamente; sui rimorsi, lì non si potrà provvedere: sui rimorsi per per i 2.300.000 italiani che sono senza lavoro, per il 12 per cento delle famiglie al di sotto della soglia di povertà, per le piccole e medie imprese che ogni giorno, a migliaia, chiudono i battenti. Su questi rimorsi noi dell'Italia dei Valori vogliamo vigilare attentamente, faremo la nostra parte e la faremo sino in fondo. Presidente, onorevoli colleghi, se l'Italia fosse una cristalleria penso che l'avreste fatta completamente a pezzi in questi giorni, tanta è stata la pesantezza, la mancanza di grazia istituzionale e la sconsideratezza con cui vi siete mossi. L'ultimo episodio è questo della fiducia che avete posto inspiegabilmente, facendoci tra l'altro un favore perché dimostrate così la vostra attuale fragilità politica, il vostro disorientamento, la vostra superficialità e ancora una volta la vostra paura ad affrontare un dibattito aperto e democratico. Sembra quasi che vi vergogniate anche voi di questo provvedimento e vogliate chiudere velocemente la pratica! Ci auguriamo che l'opinione pubblica prenda coscienza di ciò e si comporti di conseguenza. Ma questa fiducia è solo l'ultimo degli anelli di una lunga catena. Voglio ricordare l'afasia con cui avete accompagnato l'intollerabile intreccio che sta emergendo tra politica, potere dello Stato, malaffare e degrado morale: avete risposto con un decreto anticorruzione che è già scomparso dalla cronaca parlamentare, vero fumo negli occhi, per non parlare di fatti veri. E le liste cosiddette pulite sono rimaste esattamente quelle che erano e che dovevano essere, esclusi almeno coloro che sono ancora detenuti. E poi, un altro episodio: questo pasticcio delle liste. Bisogna dire con chiarezza che avete sbagliato a presentare le liste e, invece di aspettare la sentenza del TAR, avete forzato con un decreto mai visto, e che solo il grande senso dello Stato e di responsabilità del presidente Napolitano ha permesso che fosse trasformato in legge. Ma anche questo Ma anche questo non è servito a nulla e, invece di gridare ancora oggi sui giornali ai complotti e all'odio che semina la sinistra, non sarebbe stato un atteggiamento forse più responsabile ammettere gli sbagli e chiedere a tutti aiuto per rimediare e recuperare il senso di una democrazia compiuta? Con tutti questi comportamenti, in ultimo la fiducia che state ponendo, che sono frutto di un'idea arrogante e irrispettosa dell'esercizio del potere, state indebolendo la credibilità delle istituzioni democratiche e, guardate, quando la fiducia dei cittadini nella politica viene meno, non si salva nessuno, è un *boomerang* per tutti. Ieri sera il senatore Quagliariello ha paradossalmente richiamato l'etica della responsabilità;

di cui voi, anche con questa fiducia, state facendo esattamente carta straccia. Avete inaugurato l'idea che tutto sia possibile, che i diritti ed i doveri siano un impedimento e non il filo che tiene insieme la società e che regola la convivenza. Ma se manca la visione di bene comune da una parte, e saltano le regole dall'altra, la società si disgrega, colleghi! Allora, diventa il *Far west*: tutti contro tutti, la celebrazione della furbizia e del potere, i deboli e gli emarginati che finiscono fuori dal contesto sociale. Non vorrei consegnare alle mie figlie una società triste e violenta, peggiore di quella che stiamo vivendo. nel Paese, nonostante la crisi, ci siano ancora grandi energie e voglia di fare, ma così facendo non lo aiutate, lo fate andare a gambe all'aria.

quella della ripartenza, capace di un grande progetto di coesione sociale, di grandi riforme fiscali, economiche e del *welfare*. Non so, colleghi della maggioranza, che idea di Stato e di democrazia abbiate, o se ne abbiate una oltre alla difesa ad oltranza del capo; ma usciamo da questo buco nero in cui avete portato il Paese e finiamo di occuparci dei problemi di una sola persona, perché milioni di italiani aspettano che voi e noi ci occupiamo anche un po' dei loro problemi.

La Costituzione affida la garanzia dei diritti alla libera valutazione del Parlamento e al controllo di una magistratura indipendente. Nel momento in cui la voce del Parlamento viene spenta (lo abbiamo già visto con il processo breve) e si prospettano radicali riforme come quella che oggi vi accingete ad approvare, sacrificando (oltretutto con legge ordinaria) i valori della giurisdizione, una erosione, una pseudo-riforma costituzionale è già in atto, nel modo più inquietante. Oggi il Senato si appresta ad approvare con l'apposizione di due voti di fiducia - il trentesimo e il trentunesimo - la ventesima legge *ad personam*, l'ennesima legge scritta apposta per il *Premier* ed estesa ai suoi Ministri. Si tratta di un atto di prepotenza e di arroganza da parte del Governo e della maggioranza, che ormai non hanno più ritegno per raggiungere un obiettivo (il 27 marzo si profila un'altra udienza del processo Mills) e ha paura di contarsi al proprio interno. Noi avevamo preparato una serie di emendamenti su cui intendevamo confrontarci in un pubblico dibattito, quello sottoposto ad un controllo del popolo, tante volte evocato; ma la maggioranza si è sottratta per evitare che qualche emendamento potesse sfuggire al controllo e potesse essere approvato, imponendo un altro passaggio alla Camera. Non c'è alcun motivo di rischiare, ha dichiarato qualche esponente di maggioranza. Certo, qui rischia solo la Costituzione. Ma che importa? La norma che la maggioranza si accinge ad approvare è una nuova versione di una norma di procedura penale che si applica a tutti i cittadini e che, come è stato giustamente evidenziato, tutti i codici di procedura penale successivi a Torquemada hanno sempre previsto: il rinvio del processo quando l'imputato è impossibilitato a comparire L'imputato, per difendersi, ha diritto di essere presente. Se non gli è possibile perché è ammalato o perché ha avuto un incidente stradale o un problema insormontabile, non si può celebrare il processo in sua assenza. Ovviamente, si chiede al giudice di valutare se l'assenza sia dovuta ad impossibilità a comparire, in maniera da rinviare il processo senza timore che la giustizia (un valore costituzionale) venga beffata e vengano sacrificati ingiustamente i diritti delle altre parti, *in primis* le parti offese. Ciò perché l'imputato ha diritto di difendersi nel processo, ma non dal processo, comprimendo ingiustificatamente altri valori costituzionali, come invece hanno sempre fatto il Presidente del Consiglio e alcuni altri imputati celebri a lui vicini, e quindi vogliono continuare a fare, apparentemente coperti da una legge incostituzionale. Nasce la figura che è stata definita dell'iperimputato, uguale agli altri ma diverso, ossia l'imputato politico che esercita funzioni di governo (*Premier* e Ministri) per il quale il legittimo impedimento previsto dalla legge che si applica a tutti non va più bene, perché - si sostiene - la sua qualità di politico di Governo costituisce in sé e per sé un legittimo impedimento a presentarsi nei processi in cui è imputato, anche per reati comuni, anche per quelli commessi prima di assumere la carica. Un politico che abbia funzioni di governo, come il Presidente del Consiglio o un Ministro, teoricamente può andare in vacanza, alle inaugurazioni, a convegni, a manifestazioni di ogni tipo, se necessario anche utilizzando gli aerei di Stato, ma non presenziare e difendersi nel processo che lo riguarda: è legittimamente impedito e può farselo certificare dai suoi funzionari (ovvero autocertificare) in modo continuativo per diciotto Tutto ciò naturalmente è incostituzionale: che vi siano qualifiche personali e corrispondenti impegni professionali incompatibili con il processo penale e altre qualifiche e impegni che non lo sono, tranne casi da valutare volta per volta, è in evidente violazione dell'articolo 3 della Costituzione. Per esempio, perché i Ministri sì e i Sottosegretari no? perché no i presidenti delle Regioni? Forse hanno meno da fare del Ministro per le pari opportunità o dei Ministri senza portafoglio? Ma il *Premier* e i Ministri hanno davvero un'incompatibilità ontologica con il processo? prevista per un chirurgo oncologo che trascorre in ospedale il suo tempo continuativamente e da cui dipende la salvezza di vite umane? La conclusione è amara e dimostra tutta la valenza di questa tecnica di erosione della Costituzione e della democrazia: anche se così fosse, ritengono Governo e maggioranza, guadagniamo tempo fino a quando il lodo Alfano costituzionale (tra l'altro una legge di difficile elaborazione) sarà approvato. Ecco disvelata una spudorata tecnica, un rituale cui Governo e maggioranza ci sottopongono da tempo: emanare in serie leggi incostituzionali, che comunque impediscano ai tribunali italiani di processare il Presidente del Consiglio (e ora anche i suoi Ministri, qualcuno dei quali ha già qualche problema giudiziario). Quando una legge sarà giustamente dichiarata incostituzionale, ne sarà pronta subito un'altra, gridandosi contemporaneamente al complotto, e quando anche questa cadrà, ce ne sarà un'altra ed ancora un'altra; e così via, fino alla soluzione naturale del problema. La maggioranza, che non ha il coraggio di sottrarsi al voto che il *Premier* (ora ancor più spalleggiato da tutta la compagine dei Ministri, che ha diretto interesse alla normativa) le impone, sostiene che spetta solo al popolo decidere chi deve governare, e non a qualche magistrato. Considerazione assolutamente condivisibile, poiché alla magistratura compete solo di stabilire se un imputato è colpevole o meno. Ma questo non sarà più possibile, perché quando il processo riprenderà per un legittimo impedimento così configurato sarà passato troppo tempo. Ingiustizia è così fatta, la legalità sacrificata e la democrazia sempre più si indebolisce in questo Paese e muore, ignorandosi tra l'altro qualsiasi evidente conflitto di interesse. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, senatrici e senatori, l'aver posto la fiducia su un disegno di legge di iniziativa parlamentare costituisce un'assoluta anomalia nel quadro dei rapporti politici e istituzionali, anomalia sostanzialmente senza precedenti. Né il Ministro dei rapporti con il Parlamento, né il Presidente del Consiglio, assente, né il Ministro della giustizia hanno motivato questa richiesta. Si tratta di un atto di arroganza che evidenzia una grave mancanza di rispetto verso il Senato e che aumenta la sfiducia dei cittadini verso le istituzioni democratiche. Qual è, Presidente, la condizione per la quale la maggioranza e il Governo cadrebbero se non venisse approvato subito questo disegno di legge? La fiducia evita di pronunciare in questa Aula istituzionale la vera causa di questo di questo provvedimento, così come ha indicato la senatrice Adamo nel suo intervento. La fiducia ha l'obiettivo di impedire un dibattito serio e approfondito, peraltro già compresso dai tempi contingentati e di impedire, sia alla maggioranza che all'opposizione, Il Governo, tra l'altro, pone la fiducia su un atto che presenta, com'è sottolineato nella pregiudiziale di costituzionalità presentata dal Partito Democratico e illustrata dal senatore Ceccanti, evidenti elementi di costituzionalità, in violazione degli articoli 3 e 138 della Costituzione. La fiducia e questo disegno di legge, ancora una volta, evidenziano il disprezzo da parte della maggioranza e del Governo per la Costituzione, per le leggi vigenti, per le regole, per l'uguaglianza dei cittadini, per la parità di trattamento di tutti. Le regole, Presidente, non sono un inutile orpello, non sono una forma, un intralcio, ma l'essenza stessa della democrazia. Questo disegno di legge si colloca in una lunga filiera di norme (il lodo Schifani, il lodo Alfano, il processo breve e ora il legittimo impedimento) che sono state giustamente definite leggi *ad personam*, per una persona, il Presidente del Consiglio. leggi che comunque determinano delle prerogative a favore di cariche istituzionali che possono essere attribuite - è stato più volte ribadito dalla Corte costituzionale - soltanto dalla Costituzione o da una legge di rilievo costituzionale. Quando questi disegni di legge sono stati approvati e diventati legge sono stati sempre dichiarati incostituzionali. È un disegno di legge così evidentemente incostituzionale che l'articolo 2 dello stesso sente il dovere di definire questa legge come un ponte verso una normativa successiva, che prenderà Presidente, personalmente provo un senso di umiliazione democratica, un disagio vero nell'intervenire in questa Aula per esprimere queste valutazioni, perché l'assenza del Presidente del Consiglio e il silenzio di tutti gli esponenti del Governo presenti, ancora una volta, esprimono una concezione del governo come comando, come imposizione delle proprie scelte al di fuori di ogni confronto parlamentare, al di fuori del rispetto del principio della divisione e dell'equilibrio dei poteri. Ho fatto parte del Governo nazionale, del Governo regionale e dei governi locali e proprio da queste esperienze ho tratto il senso che il governare significa innanzitutto saper ascoltare, conoscere e ascoltare i punti di vista e i bisogni, valorizzare le competenze e saperi. Governare significa concertare le scelte, condividere gli obiettivi e gli strumenti attraverso i quali perseguirli, pur in presenza di visioni politiche assolutamente differenti. Questo metodo credo che sia giusto sempre, ma è giusto a maggior ragione oggi in un Paese in crisi, che ha grandissime difficoltà economiche, occupazionali e sociali, in un Paese con il debito pubblico tra i più alti del mondo che cresce nonostante i violenti tagli del ministro Tremonti su settori settori fondamentali per il futuro del Paese come la scuola e l'università. Il Governo dovrebbe proprio cercare la concertazione dei soggetti, delle parti sociali, il confronto con le forze politiche tutte, anche con quelle dell'opposizione, occupandosi in via prioritaria dei problemi del Paese. Presidente, il consenso popolare anche maggioritario e ampio non scioglie chi lo ha ricevuto dal rispetto delle leggi, così come invece pensa e troppo spesso dichiara il Presidente del Consiglio. Governare non è comandare, non è porsi arbitrariamente al di fuori delle leggi o avere il diritto di cambiarle a proprio vantaggio, come dimostrano da ultimo

che l'ideologia del "comando per fare e risolvere i problemi", del «ci penso io, non vi preoccupate», costantemente richiamata dal Presidente del Consiglio, sia un'ideologia falsa, falsa, perché i problemi non sono niente affatto risolti e perché cerca di camuffare l'idea del comando come privilegio di pochissimi, a danno di tutti. Penso che i cittadini ormai se ne siano accorti e quel consenso tante volte citato come legittimazione dal Presidente del Consiglio già dalle prossime elezioni vedrà una significativa diminuzione.

è palesemente contrario ai princìpi generali dell'ordinamento e allo Stato di diritto. Mi soffermerò nel mio intervento su alcuni aspetti che riteniamo più gravi dell'articolo 1. Sotto il profilo costituzionale, è assolutamente inopportuno concedere anche ai Ministri il diritto a non presentarsi in udienza. proprio negli ambienti della maggioranza - che «il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Presidente della Repubblica esercitano le loro funzioni tipiche soprattutto come organo individuale e non come organo collegiale». A tal proposito, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 262 del 2009, ha ribadito come risultasse eventualmente di «apprezzabile interesse» assicurare «il sereno svolgimento delle rilevanti funzioni che ineriscono a quelle cariche»; quelle cariche cioè (e non altre) menzionate nella legge Schifani prima e nella legge Alfano dopo, leggi dichiarate incostituzionali nel loro complesso. Non a caso l'articolo 205 del codice di procedura penale, trattando della «Assunzione della testimonianza del Presidente della Repubblica e di grandi ufficiali dello Stato», menziona solo e soltanto il Presidente del Consiglio dei ministri, e non anche i singoli Ministri. Del tutto irragionevole è la norma per cui i Ministri ed il Presidente del Consiglio, in virtù del concomitante esercizio di una o più delle attribuzioni previste dalle leggi e dai regolamenti e, comunque, attribuzioni connesse alle relative attività preparatorie consequenziali, sarebbero legittimamente impediti a comparire davanti ad un tribunale ordinario, mentre tale impedimento non sussisterebbe e non sarebbe invocabile per i reati ministeriali. La medesima circostanza produce dunque - questo è il senso - effetti diversi a seconda del tribunale davanti a cui si celebra l'udienza e del reato per cui si procede. Avendo la legge costituzionale disciplinato i reati ministeriali, ben avrebbe potuto, dal punto di vista formale (articolo 138 della Costituzione) se non sostanziale (articolo 3 della Costituzione), individuare una sorta di legittimo impedimento a comparire.

Oltre alla indeterminatezza oggettiva del comma 2, che equipara Ministri senza portafoglio e Ministri con portafoglio, emerge con tutta evidenza la discrezionalità assoluta in merito alla decisione dell'utilizzo del legittimo impedimento ad ad appannaggio dell'attuale presidente del Consiglio, onorevole Berlusconi, in considerazione del fatto che l'istituto si estende ai Ministri ma è di fatto il Presidente del Consiglio che ne ha bisogno. Il Presidente del Consiglio, com'è noto, propone - ai sensi dell'articolo 92, primo comma, della Costituzione - la nomina dei Ministri e potrebbe - in via teorica - proporre al Presidente della Repubblica la nomina di un Ministro (magari senza portafoglio) imputato in un procedimento penale, proprio per conferirgli l'immunità processuale attraverso il legittimo impedimento di cui al presente provvedimento. E non si comprende perché un diverso trattamento non sia riservato ai reati commessi anteriormente all'assunzione della carica di Governo, dei quali chi accetta la nomina a Ministro è ben consapevole. L'istituto del legittimo impedimento - così come è delineato dal disegno di legge in oggetto - è preso a pretesto ed irragionevolmente forzato fino a farne una vera e propria «prerogativa oggettiva e soggettiva» delle cariche ricoperte dai suddetti membri di Governo. Del fatto che - come si è cercato di dimostrare - una simile prerogativa non con legge ordinaria appare consapevole lo stesso disegno di legge all'articolo 2, che quindi indirettamente dimostra l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'articolo 1. Come affermato da illustri costituzionalisti in audizione in Commissione giustizia alla Camera dei deputati, si tratta «non di una legittima disciplina del processo, rimessa al legislatore ordinario, ma di una forma di deroga al normale esercizio della funzione giurisdizionale, che solo il legislatore costituzionale potrebbe eventualmente stabilire. L'impedimento legittimo è, infatti, per sua natura, qualcosa di puntuale e concretamente localizzato nel tempo: una presunzione *ex lege* assoluta di impedimento "continuativo" per un lungo periodo di tempo equivarrebbe ad una norma di *status* derogatoria, cioè appunto ad una prerogativa». Dunque, la prospettiva introdotta dal disegno di legge in oggetto, rinunciando a qualsiasi collegamento oggettivo con le funzioni esercitate, risulta differenziarsi sul piano sistematico da tutti gli altri casi previsti nel nostro ordinamento. L'immunità è uno strumento per assicurare l'autonomia dall'organo costituzionale, non il privilegio dell'investitura. Il *vulnus* alla democrazia inferto oggi con questo provvedimento e con questa fiducia dimostra che, invece, quello che vuole questa maggioranza è soltanto privilegiare pochi a discapito di molti. Signor Presidente, in verità - come hanno fatto molti colleghi - pensavo di articolare questo mio intervento su una riflessione tecnico-giuridica che avesse ad oggetto soprattutto la clamorosa congerie di profili di illegittimità costituzionale che presenta il provvedimento che vi accingete ad approvare

che si aggira per le aule universitarie e fra i corsi di diritto costituzionale. Sembra quasi che sia stato redatto da qualcuno che desiderava proporre agli studenti del corso di diritto costituzionale al primo anno di università un piccolo o grande - orrore giuridico nel quale costoro, con il bisturi della matricola, potessero esercitarsi ad individuare le molteplici ragioni di contrarietà alle norme della Costituzione, e in particolare agli articoli 3,

lo ripeto, e concludo sul tema dei profili di incostituzionalità, che in realtà appaiono non interessare nessuno - che questo provvedimento presenti una caratteristica che lo rende unico nella storia della legislazione, unico per la sua straordinaria autoreferenziale abnormità, perché contiene in se stesso l'esplicita certificazione della sua incostituzionalità. Mi riferisco al fatto di dire che un provvedimento legislativo viene adottato in attesa che, fra diciotto mesi, intervenga il provvedimento legislativo che effettivamente può disciplinare la materia in ossequio alla gerarchia delle fonti, cioè la legge costituzionale. Ebbene, è corrispondente - questa sì - ad una certificazione diversa da quella che l'impiegato della Presidenza del Consiglio dei ministri dovrà dare invece al Presidente del Consiglio perché possa sottrarsi, cioè fuggire alla giurisdizione, così come oggi fugge non al giudizio dell'Aula, ma alla naturale sede del confronto democratico. Interroghiamoci su quante volte abbiamo avuto a seconda dei punti di vista - il piacere o il dispiacere di vedere in quest'Aula il Presidente del Consiglio. È qualcosa che ha a che fare con un minimo di fisiologia della vita democratica il fatto che il capo della maggioranza si rifiuti sistematicamente di venire a fare il - mi permetta, signor Presidente - che lo faccia anche in maniera sprezzante nei confronti della seconda carica dello Stato, da lei rappresentata, non ritenendo cioè neanche di fornire un'indicazione su ciò che gli impedisce di fare il suo dovere democratico, su ciò che gli impedisce di venire ad affrontare, a viso aperto, i rappresentanti del popolo, che troppo spesso gli piace evocare a sproposito, nel momento in cui giunge a compimento un disegno che viene da lontano, quello della distorsione del sistema normativo e legislativo per fini personali. Cito soltanto un rapido elenco, prima di dire ancora solo alcune cose ed avviarmi alla conclusione, con anticipo, perché amo le regole e amo rispettare i termini: legge sulle rogatorie internazionali, 2001; depenalizzazione del falso in bilancio, 2002; legge Cirami, 2002, lodo che porta il suo nome, signor Presidente, 2003; decreto-legge salva Rete 4, 2003; legge che prende il nome dal capogruppo della maggioranza in Aula, 2004; condono edilizio nelle aree protette; legge ex Cirielli; legge Pecorella; lodo che prende il nome dal dal Ministro della giustizia che ci ha fatto l'onore di essere qui presente per un po' (e che poi, naturalmente, in base ad una gerarchia di impegni, ha dovuto allontanarsi); legge Tremonti-*bis*, decreto-legge salva calcio; condono tombale; incentivo per l'acquisto del *decoder*; riordino per la previdenza complementare; decreto-legge anticrisi. recentissime spiacevoli ulteriori vicende normative, che culminano in questa che, oltre ad essere una vicenda normativa in sé, è una metafora di uno stato del Paese: stato del Paese che, purtroppo, è possibile registrare da molti inquietanti fattori. Ve ne voglio raccontare uno che forse ai più è sfuggito. Può sembrare una piccola cosa, un indizio, invece è significativamente enorme. Qualche settimana fa era in televisione il sottosegretario Bertolaso, una sorta di creatura mitologica, perché egli assomma in sé - anche in questo abbiamo interessanti esperimenti di genetica costituzionale - il ruolo di alto funzionario dello Stato e, al tempo stesso, di soggetto con incarico politico in quanto sottosegretario, per l'appunto. Nel momento in cui si parlava della tragica, triste, spaventosa vicenda dell'indagine in corso che ha portato all'inizio del disvelamento di un grumo di malaffare

una serie di conversazioni che riguardavano lui e la sua struttura, i carabinieri non l'avessero avvertito. Guardate, questa è una metafora. Questo piccolo fatto è una metafora, perché Bertolaso non stava facendo finta, come spesso capita di verificare.

per cui se i carabinieri ascoltano una intercettazione nella quale si parla di reati non vanno dal funzionario pubblico o dal Sottosegretario o dal "superuomo" della Protezione civile - uomo le cui doti tecniche credo non siano in discussione - a dirgli che c'è un certo problema, e chi se ne importa se c'è l'indagine, se ci sono i magistrati e se ci sono le regole. Le regole ci sono anche se la sistematica "truffa delle etichette" che il Governo e la maggioranza portano avanti con ostinata determinazione

se presente in questa Aula è una parola un po' grossa - ricorderà chi adoperò questa espressione e, quindi, la nobiltà della citazione. Ma - ripeto - non parlo di truffa delle etichette a cuor leggero.

del corpo. Metaforicamente, io parlo in questo caso di impedimento - quello che si chiede di approvare in quest'Aula - come drammatica, definitiva minorazione democratica permanente di chi sfortunatamente oggi ci governa.

Capisco che lei ha sostenuto che la sostanza è quello che conta, e non la forma, ma mi chiedo se, qualora andassi a fare questo mio intervento seduto al posto del Presidente del Consiglio dei ministri o in braccio a lei, lei me lo permetterebbe. Penso Penso di no, ma vedo che con distrazione fa finta di niente, e me ne dispiace, perché penso che anche sotto questo profilo si debba cercare di tutelare le prerogative del Parlamento.

né sull'assurdità politica di questo dibattito né sulla incostituzionalità del testo che esaminiamo, anche perché sono tutte riassumibili nel fatto che l'impedimento, così come congegnato nella norma, si trasforma in un'immunità temporanea, riconosciuta in ragione della funzione esercitata, e quindi nulla distingue nella sostanza questo istituto da quello della sospensione dei processi per le alte cariche dello Stato stabilito con il lodo Alfano bocciato dalla Corte costituzionale per violazione del principio secondo cui tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge penale. Non volendo entrare nel merito di queste argomentazioni, faccio alcune considerazioni partendo dai numeri. Potrei citare il numero delle questioni di fiducia poste dall'inizio di questa legislatura: oggi assisteremo alla trentesima e alla trentunesima. Avevo perso il conto, ma quello che invece ho ben chiaro stampato nella mente è la considerazione che ha questo Esecutivo del Parlamento, proprio in ragione del paradigma di queste fiducie: nulla di più che un necessario intralcio causato dalla democrazia. Tanto basterebbe che votassero i Capigruppo, così come sostiene il Capo di questo Esecutivo. Potrei citare il numero delle leggi *ad personam* di questa malconcia seconda Repubblica, riferendo quel *ad personam* nel senso di in funzione del Presidente del Consiglio dei ministri.

a cui se ne devono aggiungere 11 che potremmo definire *lato sensu* abortite, nel senso che sono di diverse fattispecie: alcune progettate,

ce ne sono anche altre 16 *ad personam*, nel senso che sono fatte per altre persone, o contro qualche altra persona: una per tutte, quella concepita contro il procuratore Caselli.

invece ci stupiamo, perché questo è un comportamento senza ritegno e temiamo che si possa sempre riuscire a vedere qualcosa di peggio,

se avremo tempo per tornare a parlare anche di questa nuova sciagura. Tornando al disegno di legge al nostro esame, nella *vulgata* è passato come legittimo impedimento, anche se di legittimo non ha assolutamente nulla, se non la testimonianza della capacità del centrodestra di utilizzare i mezzi informativi asserviti per far passare all'esterno il messaggio che si ritiene necessario, così come quando come quando la maggioranza continua a definirci - noi che abbiamo espulso la sinistra radicale - la sinistra, e non il centrosinistra, e loro - che nascono dalla fusione con un partito postfascista - a definirsi centrodestra, invece che destra.

di fuggire dalle sue responsabilità pregresse col pretesto dei doveri del suo attuale ufficio. È in questo contrasto, in questo non senso tra il pregresso e l'attuale, che sta tutto il limite e la pochezza di questo provvedimento. E non si venga a dire, come è stato fatto anche in Commissione, che questo è un ponte tibetano proteso verso la legge costituzionale che, in futuro, dovrà proteggere le cosiddette alte cariche istituzionali dai procedimenti giudiziari a loro carico: carico: oltre ad introdurre la buffa fattispecie della legge ponte, su cui si è ben soffermato il collega Ceccanti, in realtà, ed in modo disperato, qui si persegue solo la logica del male minore.

Guardate, la logica del male minore non può essere accettata, perché, come ricordava Paolo Sylos Labini, il male minore non esiste: è solo una porta aperta verso il prossimo male peggiore. Ciò che si intravede all'orizzonte di questo provvedimento è il rischio dello stravolgimento degli equilibri fra i poteri dello Stato. É la politica nella sua accezione deteriore che rafforza il suo potere indebolendo gli organi di garanzia e i controlli. È un *climax* crescente, che parte dai condoni per gli evasori fiscali, passa a quelli per i devastatori del paesaggio ed arriva allo scudo fiscale per i patrimoni illegali, in un'orgia di potere che rende lecito l'illecito sotto il crisma del consenso avuto dal popolo, ma non esercitato nelle forme e nei limiti della Costituzione. Con questa legge la bilancia della giustizia viene falsificata ufficialmente e formalmente dalla maggioranza del Senato.

«se obbediamo solo alle regole che riteniamo giuste e ragionevoli, allora qualsiasi regola cessa di avere valore, perché non esiste una regola giusta e ragionevole per tutti. E se ci interessa solo il nostro tornaconto personale, troveremo sempre una giustificazione per definire ingiusta una regola restrittiva. Si comincia con un trucco astuto e si finisce con l'anarchia e la catastrofe, così, anche per lo scaltro autore del trucco, dal momento che nemmeno lui sopravviverà al crollo della società». Asimov era uno scrittore di fantascienza, ma il nostro Paese purtroppo tutto ciò rischia di doverlo vivere nella tragica realtà. il Gruppo Italia dei Valori sta facendo una protesta gandhiana, pacifica e non violenta,

Mentre noi discutiamo sul legittimo impedimento, che stasera vi approverete dopo aver posto il trentesimo voto di fiducia ed aver sequestrato le prerogative delle Camere piegandole agli esclusivi interessi di pochi, il Paese reale - non quello rappresentato dalle veline dei TG TG lette da giornalisti compiacenti che ogni sera cercano di rassicurarci sugli effetti della gravissima crisi, che sarebbe finita,

al lavoro egregio della magistratura, alla quale volete mettere il bavaglio) e ad una tenuta dei redditi delle famiglie messa a dura prova. I dati, non quelli inventati dalle opposizioni, ma quelli delle statistiche ufficiali, parlano chiaro:

per cento, con un aumento di circa 38,2 miliardi di euro; per la prima volta dal 1991, il saldo primario è negativo. Questi sono i dati

di circa 130.000 su 3,5 milioni di mutuatari, di 20.000 procedure avviate nel 2009. Insomma, i pignoramenti farebbero sparire una città media come Monza. Questi dati, oltre a dimostrare che la crisi non è ancora alle spalle, sono un duro monito sia per il Governo, che dovrebbe intervenire per adottare politiche economiche di contenimento e di sussidio per le famiglie, che per le banche, che dopo aver prodotto una crisi senza precedenti strozzano i consumatori con una fortissima restrizione del credito, tassi troppo elevati e condizioni capestro. Le banche continuano a fare il bello e il cattivo tempo, come dimostra l'ultima infornata di nomine, per ridisegnare gli assetti del cosiddetto capitalismo aduso a capitalizzare i profitti e a socializzare le perdite. L'amministratore delegato della Cassa depositi e

soffre una crisi senza precedenti, voi, signori della maggioranza, sequestrate il Parlamento per garantire l'immunità a pochi, senza affrontare nessuna delle questioni che ho ricordato. Per tale

Signor Presidente, vorrei fare una premessa a questo mio intervento.

Fatta questa premessa, qual è, a mio avviso, il problema principale di questa richiesta di fiducia? La concezione del potere come impunità. Lo hanno detto molti colleghi che hanno parlato prima di me. Ricordo l'egregio intervento del senatore Procacci: avete un'idea del consenso quale fatto superiore alle regole e allo Stato. Dice ancora: guardate che questa è un'idea eversiva, riflettete.

«La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione». Anche la seconda parte del comma va tenuta presente. C'è una concezione del potere come impunità: è evidente rispetto alla questione delle regole violate sulla presentazione delle liste. Leggo oggi sulla stampa che la maggioranza, il Presidente del Consiglio stesso sembrano dire: c'è un disegno contro di noi; è un sopruso; è colpa della magistratura, dell'opposizione, della sinistra. C'era un tempo dato - le ore 12 del 27 febbraio - per presentare le liste e le firme. Guardate, è l'esperienza che in Italia

si insegna che non si deve barare, che è bello giocare se si rispettano le regole. Tra l'altro, sembrava che anche negli insegnamenti che volevate portare nella scuola (l'idea del grembiule, del 5 in condotta) vi fosse la

rimanda l'esame e decide di partecipare la volta successiva. È l'esperienza che fa l'automobilista: c'è un codice della strada che deve rispettare, altrimenti vi è la contravvenzione. È l'esperienza che fa l'imprenditore che decide di presentarsi ad una gara: comunque, sa che quello è l'orario, quello il momento ed il punto, altrimenti la sua proposta verrà esclusa. Allora, perché per chi fa politica, per la maggioranza che fa politica e, quindi, è la prima a fare le regole, queste non devono valere? Perché la politica può barare? C'è una concezione del potere come impunità anche in questa vicenda che stiamo vivendo, a cui il Paese guarda con particolare angoscia e che fa aumentare il disprezzo del Paese nei confronti della politica a causa degli scandali e della corruzione.

C'è una concezione del potere come impunità anche in questa richiesta di fiducia su una legge di iniziativa parlamentare (lo hanno ricordato i colleghi: non è mai avvenuto che ancora una volta mette in luce come una legge elettorale che di fatto decide già chi verrà eletto, secondo l'ordine di lista, rende il Parlamento molto meno forte nella capacità di rapportarsi come forza a sé stante nei confronti del Governo.

Rispetto a tali considerazioni, vorrei riferirmi al richiamo all'etica della responsabilità che è stato fatto ieri dal senatore Quagliariello

del tempo che in questi due anni abbiamo dedicato ai problemi giudiziari del Presidente del Consiglio. Voi siete molto abili nel fare questo ribaltamento: l'opposizione, ossessionata da Berlusconi, parla solo dei problemi giudiziari. No, avremmo voluto, in questi due anni, parlare molto di più di questa crisi terribile che attanaglia il Paese, di quello che potremmo fare per evitare che i lavoratori vadano sui tetti, di quello che potremmo fare per migliorare tutte le situazioni che sappiamo non andare, anche la giustizia,

abbiamo opinioni diverse su alcuni punti ma ci sono questioni su cui, riportando ad un livello normale la politica di questo Paese, è possibile un rispetto reciproco e su di esso costruire per il Paese. Era iniziata così questa legislatura, e c'era una grande attesa da parte dei cittadini che la politica riuscisse a fare quel salto, che non fosse solo sempre gazzarra e solo contrapposizione. Ma poi è colpa dell'opposizione se è cambiato il tono, il clima di questa legislatura? No, è colpa del fatto che si sono intensificate le udienze per il processo Mills e per il processo

una legge per tutti, che comunque diventasse di fatto la negazione stessa della giustizia, e quindi il bloccaprocessi, o una legge *ad personam*, e quindi il lodo Alfano, in modo tale da avere una sorta di pistola puntata sul Parlamento. Come dire: o

parlamentare su problemi personali legati alla giustizia non ha dimostrato né forza né capacità di governo. Questa è una prova di debolezza, non una prova di forza. Signor Presidente, colleghi, una brevissima risposta all'amico e collega Mauro Marino. Penso abbia sbagliato ad evocare l'idea del bivacco: questo non è un bivacco, ma una manifestazione molto tranquilla e silenziosa di protesta. Inoltre, il richiamo al bivacco di manipoli mi sembra storicamente fuori causa, perché lì si trattava di un potere abietto che inventava il bivacco di manipoli dentro un'Aula parlamentare, qui siamo l'opposizione, quindi non possiamo in alcun modo minare la salute di quest'Aula. Lo hanno detto già molti colleghi: la legge è incostituzionale e l'avvilimento crescente è dovuto al fatto che c'è anche un impedimento al dibattito parlamentare. L'impedimento al dibattito parlamentare va preso sul serio: ci sono menti che sono state

degli effetti dell'anomalia italiana. Siamo vincolati, senza volerlo, a questa storia infinita che ripete continuamente episodi tutti simili l'uno all'altro e tutti peggiori l'uno rispetto all'altro, con un crescendo inarrestabile. Si dice che c'è lo scontro tra la magistratura e il potere politico, e si dimentica che il potere politico ha un saldo controllo sull'informazione. Questa è l'anomalia italiana: lo scontro tra magistratura e potere politico e saldo controllo del potere politico sull'informazione. Le due cose hanno un rapporto simmetrico: solo con il saldo controllo sull'informazione si può sostenere l'invenzione di uno scontro tra la magistratura e il potere politico. La storia delle ultime legislature e la storia dei processi dimostrano, ad abbondanza, che i motivi dell'azione giudiziaria erano tutt'altro che inventati, che i processi sono stati evitati con la modifica forzosa della legge che li riguarda.

lo dimostrano le stesse leggi *ad personam* che insistono sul loro ridimensionamento; ma i soldi transitati dalle aziende del Presidente del Consiglio a Craxi per premiarlo dell'intervento sulle leggi relative alle reti Tv sono una cosa conclamata. L'acquisizione di Mondadori con i soldi transitati attraverso i conti di Previti sono un'altra cosa conclamata. Come si fa a dire che c'è uno scontro tra politica e magistratura? C'è semplicemente da parte della magistratura l'accertamento e, in qualche caso, il faticoso perseguimento di di processi in merito. Il possesso e il controllo dei mezzi di comunicazione garantiscono una falsificazione sistematica dei fatti e l'inquinamento della vita pubblica. Per esempio, si racconta la favola, la leggenda metropolitana per cui saremmo in un clima di guerra civile. Basta mettere il naso fuori di quest'Aula per vedere come i difficilissimi problemi sociali del popolo italiano, dell'economia, della disoccupazione, del lavoro precario, del lavoro finanche gratuito, della mancanza di nerbo dell'azione economica della società non si traducono mai in disordine sociale. Nessuno si approfitta della difficoltà della situazione per fare blocchi stradali, buttare bombe, aggredire i nemici. Dov'è la guerra civile? guerra civile? La guerra civile sta solo in un fatto: c'è un'azione dell'anomalia italiana che insuffla irresistibilmente veleno qui L'unica guerra civile è quella portata dall'anomalia italiana con il veleno dentro le istituzioni e con l'inquinamento della politica alle sue radici. Non c'è un'altra guerra civile. Con lo strumento in mano del controllo e del possesso dei mezzi di comunicazione si contrabbanda l'ultima cosa impossibile: l'elezione diretta dell'eletto. «Io sono eletto direttamente dal popolo». Ma mai balla più colossale è stata sostenuta dentro la società italiana! C'è perfino un analfabetismo costituzionale, l'ignoranza delle leggi. Dove sarebbe la legge apposita che ha stabilito che il popolo italiano vota un Presidente eletto direttamente dal popolo? C'è un solo piccolo e miserabile trucco iconografico nel modulo con cui si vota, un trucco che forse metà degli elettori non ha nemmeno visto: l'indicazione del *Premier*. Cari colleghi, l'indicazione del *Premier* non è l'elezione diretta del Presidente del Consiglio. La banalità della televisione si accoppia all'ignoranza, e ne vediamo le ulteriori conseguenze: il cosiddetto eletto direttamente dal popolo si permette addirittura di minacciare il Quirinale, il Presidente della Repubblica. Non è un mistero per nessuno: lo hanno scritto giornalisti al di sopra di ogni sospetto e, persino, Bruno Vespa, l'insospettabile, ha scritto di una notte tumultuosa nella quale il Presidente della Repubblica è stato sottoposto a pressioni inenarrabili.

qualche mese di silenzio di tutti su questo argomento, che tutti consideravamo demolito dall'avventura delle *escort*, degli scandali, di tutto il resto che non sto qui a richiamare, l'onorevole Franceschini di nuovo teme la possibilità di una prospettiva che questo finto eletto direttamente dal popolo possa aspirare addirittura a salire al Quirinale. Assisteremmo all'ignominia massima della Repubblica italiana: chi ha svuotato e chi svuota la Costituzione tutti i giorni seduto sullo scanno di chi invece deve garantire la sanità della Costituzione. Chi si opporrà a tutto questo? Non solo noi, non solo l'opposizione parlamentare, ma anche il popolo senza guerra civile: il popolo tranquillo, saggio, che affronta queste difficoltà economiche, le difficoltà della vita quotidiana, misurandosi con le iniziative di lotta pratiche, con la capacità di rivendicazione, con l'inventiva creativa e senza nessuna violenza. Questo popolo saggio impedirà questa ignominia della Repubblica italiana.

Signor Presidente, siccome il senatore Lannutti ha evocato la nonviolenza gandhiana e siccome io ammiro e stimo il suo eccellente lavoro parlamentare, mi corre l'obbligo di spiegare un minimo - mi perdonerà la senatrice Carlino che dice che faccio lezioni! - cos'è la nonviolenza gandhiana: non perché io ne sia depositario, ma perché sono quindici anni che cerco di praticarla quotidianamente.

il terzo atto è l'affermazione di coscienza attraverso tutta una serie di ulteriori strumenti, che vanno dallo sciopero della fame allo sciopero della chiacchiera, dallo sciopero della sete allo sciopero di tante altre situazioni. Oggi noi non abbiamo assistito assolutamente a niente di tutto questo. Non lo dico perché ci sia da dare lezioni. Credo che il problema aperto con questa discesa e seduta nell'emiciclo resti ancora aperto, visto e considerato che i senatori Questori avranno negoziato non so che cosa e il risultato è che non si è mosso nessuno, ma sono usciti i senatori Questori dall'Aula. Questo credo che dovrà rimanere agli atti come un dubbio, sul quale ci aspettiamo un decreto interpretativo in merito ai tre articoli che non sono stati violati del nostro Regolamento; ma sicuramente la questione è rimasta aperta, cioè è stato tirato un sassolino in uno stagno enorme che caratterizza ormai i lavori di tutti noi. Sono però prontissimo ad essere stupito, sperando che chi si è messo a sedere per terra poi rimanga lì quando fra poco usciremo dall'Aula, e che magari lo ritroveremo sdraiato e affamato quando torneremo alle ore 15. **Mozioni